In data 14 novembre 2008, il professor Giovanni Maria Flick ha inviato la seguente lettera:

con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149, recante disposizioni urgenti per assicurare adempimenti comunitari in materia di giochi***

Signor Presidente, onorevoli colleghi, questa mattina si è svolto un dibattito molto proficuo su questo Atto Senato, significativo e importante; pertanto, delle osservazioni devono essere pur fatte.

di difficile lettura, perché vi sono anche sovrapposizioni di norme, di norme, europee con norme del nostro Stato che forse ritardano l'*iter* legislativo di questo provvedimento. Devo dire che, nonostante queste difficili interpretazioni, mettere ordine in questo settore non è misura semplice né realizzabile solo con questo provvedimento legislativo. Ritengo che la trasparenza sia necessaria nel settore dei giochi perché, come tutti sappiamo, in Italia

Stupisce un po' l'atteggiamento dell'opposizione, perché realmente il decreto è stato utilizzato per far fronte ad esigenze di necessità e urgenza, derivanti da problematiche

era ormai da considerare assolutamente non più rinviabile. Quindi, il Governo è dovuto intervenire con logiche di decretazione d'urgenza, utilizzando questo strumento proprio con l'obiettivo, che è stato posto anche dall'opposizione, di di riuscire a rendere ancora più chiara la questione della liceità del gioco, a rendere più chiari alcuni aspetti che non si sarebbero non si sarebbero potuti affrontare se non con questo strumento. È chiaro che l'obiettivo del Governo non era risolvere tutte le questioni relative alla materia del gioco, che sono molte e che dovranno essere affrontate: qui rinviamo ad altri strumenti, in particolar modo al disegno di legge che consentirà un adeguato dibattito del Parlamento, ma anche ovviamente alla possibilità penso - di poter riprendere in uno spirito diverso, anche di confronto con l'opposizione, così come manifestato alla Camera, alcune grandi questioni. Vorrei ricordare sommessamente all'opposizione che parte del testo è stata abrogata alla Camera proprio per richiesta dell'opposizione e andava nel senso di regolamentare in modo efficace il tema della raccolta a distanza del gioco *on line*, che è un tema che oggi pone serie problematiche relativamente al confine tra ciò che è gioco lecito e ciò che è gioco illecito e che non dà tutele adeguate, in particolar modo ai soggetti deboli, ai minori e a tutti coloro che possono, attraverso Internet, giocare su portali che non sono attualmente considerati gioco lecito per lo Stato italiano. Quindi: recupero di evasione, recupero di legalità, contrasto a tutta l'attività criminale che ruota intorno al gioco illecito. Nonostante questo e le dichiarazioni che sono state fatte in quest'Aula, è stato richiesto al Governo di eliminare buona parte del testo che era inserito all'interno del decreto; di intervenire con logiche di urgenza su alcune questioni, dall'altra si è chiesto al Governo (e si è ottenuto) di eliminare parti significative del testo. da parte dell'opposizione ci sia un clima migliore per il prosieguo dei nostri lavori, ma soprattutto per i futuri provvedimenti, per affrontare le questioni che sono state poste in quest'Aula e che ovviamente stanno a cuore al Governo. Alcune parti di testo che sono state inserite rispondono a richieste dell'opposizione, non a richieste della maggioranza, quindi posso ribadire che la disponibilità da parte del Governo al dialogo è piena. Dovremo poi fare i conti, come sempre, con i tempi di conversione di un decreto, che ovviamente non farà giustizia di tutti i temi che riguardano oggi le inefficienze del sistema del gioco lecito, ma che comunque verranno ripresi in provvedimenti futuri.

Innanzitutto, la raccolta delle scommesse su eventi sportivi ippici viene attualmente operata, in Italia, attraverso una rete di negozi (le agenzie di scommesse) gestiti da soggetti privati in regime di concessione con l'Amministrazione pubblica. Alla fine degli anni Novanta la rete di queste agenzie di scommesse ippiche risultava stabilizzata, sull'intero territorio, in 329 unità. Entrata in vigore la legge n. 662 del 1996 (la legge finanziaria 1997), è stato previsto un progressivo ampliamento della rete delle agenzie di scommesse ippiche e, contestualmente, una apertura alle regole della selezione concorrenziale dei soggetti che avrebbero operato, in regime di concessione, quali gestori delle agenzie in questione. Gli aggiudicatari delle concessioni in tal modo attribuite avrebbero avuto titolo ad un rapporto della durata di sei anni. All'epoca, l'ampliamento della rete fu stabilito in complessive 1.000 agenzie ippiche sul territorio. Repubblica n. 169 del 1998 trattava del caso delle 329 agenzie ippiche storiche che - pensate un po' - furono attribuite, all'epoca *intuitu personae*: cioè, aveva deciso, secondo logiche di assoluta discrezionalità, l'Amministrazione dei monopoli. Anch'esse avrebbero dovuto essere messe a gara nel rispetto dei principi del regolamento governativo e riattribuite, all'esito della procedura concorrenziale, quale quota parte delle 1.000 agenzie. La gara fu espletata nel 2000 e, all'esito, vennero attribuite 671 agenzie di scommesse ippiche; non così, invece, per le 329 agenzie ippiche storiche, che hanno continuato ad operare, immutate soggettivamente nel tempo, fino ad oggi. La Commissione europea - ecco, colleghi, che risulta strana la presa di posizione attorno alla straordinarietà del Governo - ha sottolineato immediatamente l'anomalia di questa situazione richiamando il Governo, dal 2000 ad oggi, ad un'applicazione puntuale delle regole di concorrenza. È ricorsa, quindi, alla Corte di giustizia la quale, il 13 settembre 2007, ha dichiarato l'illegittimità comunitaria della condotta tenuta al riguardo e conseguentemente stabilito che l'Italia avrebbe dovuto rimuovere

sportive; 250 concessionari che possono vendere solo scommesse ippiche. Già la gara del 2006, dunque, aveva determinato una mancanza di successo in particolar modo per la gestione della rete esclusivamente legata alle agenzie ippiche. Non può non convenirsi sul fatto che nel tempo, per stratificazioni giuridiche successive, la situazione della rete di raccolta delle scommesse sportive ovvero ippiche ovvero di entrambe

Il Governo si è fatto carico di presentare in questo decreto un progetto più ampio, che noi consideriamo più efficiente e speriamo più efficace: innanzitutto della frammentazione della rete di raccolta delle scommesse sia sportive sia ippiche (questione che è di particolare interesse), traendo peraltro spunto da una constatazione di fatto, cioè che buona parte dei concessionari per la raccolta di un tipo di scommessa in realtà già raccolgono anche l'altro tipo di scommessa e che, fra tutti, solo i concessionari che vendono esclusivamente la scommessa ippica soffrono molto la crisi di raccolta indotta dalla pochezza della loro offerta ai giocatori. Una crisi che ovviamente - com'è stato sottolineato dai colleghi - si è ripercossa negativamente sulla filiera agricola del cavallo da corsa. Per questo motivo, il Governo, attraverso questo provvedimento, risolto o intende risolvere alcune questioni: prima di tutto, l'esaurimento al 31 gennaio 2009, e conseguente revoca, delle 329 agenzie ippiche storiche; l'avvio, nel frattempo, di una procedura di gara volta ad attribuire concessioni per la raccolta contestuale ed in un medesimo esercizio di scommesse sia sportive sia ippiche, per superare così la dicotomia consentita dalla cosiddetta legge Bersani, che - come sopra illustrato - solo in 40 casi ha consentito l'attivazione di esercizi di vendita "completi" dal punto di vista del prodotto di gioco costituito da scommesse; scommesse; la garanzia che la gara sia effettiva in termini di concorrenza e selezione: la gara è per un numero definito di concessioni, fonda sulla tecnica dell'offerta a rialzo rispetto ad una soglia predefinita e non può non essere competitiva, visto che solo le offerte che si gradueranno per importo maggiore potranno vedersi aggiudicate e, finito il numero delle concessioni messe a gara, le offerte più basse rimarranno insoddisfatte; l'aspetto più importante, colleghi, cioè l'apertura della gara a soggetti, nazionali o comunitari, i quali possono versare nella condizione sia di non avere ancora, in Italia, alcun tipo di concessione per la raccolta di scommesse, sia, all'opposto, di essere già concessionari Grazie, sia, all'opposto, di essere già concessionari ad altro titolo della raccolta di scommesse su base sportiva ovvero ippica. secondo novero non possono ovviamente rientrare i titolari delle 329 concessioni storiche per la raccolta di scommesse ippiche, per il semplice fatto che esse sono in scadenza e risulteranno revocate di fatto prima dell'esaurimento della gara. possibilità si giustifica con il fatto che rientra nel progetto innovativo dell'Amministrazione dei monopoli di superare una volta per tutte la dicotomia ed asimmetria numerica fra punti di raccolta di scommesse ippiche e punti di raccolta di scommesse sportive: in futuro, dunque, esisteranno solo

alla gara, possano completare il titolo di concessione già conseguito, risultando, di conseguenza, legittimati a vendere un qualunque tipo di scommessa. Coessenziale a quest'ultima esigenza è tuttavia quella - giustificata da ragioni di equità, rispettose del principio costituzionale di parità di trattamento di riconoscere almeno un vantaggio economico al futuro aggiudicatario, che tuttavia sia già concessionario ad altro titolo (magari per essere divenuto tale di recente, investendo risorse economiche nella gara bandita nel 2006,

dovranno "restituire" le concessioni in essere nel momento stesso in cui sottoscriveranno le convenzioni accessive alle nuove concessioni. Aggiungo che l'Europa ha appena prescritto in maniera puntuale che le concessioni decadano entro il 31 gennaio 2009, quindi siamo in una condizione di sostanziale emergenza per il settore. La scadenza delle concessioni che si attribuiranno coinciderà il 30 giugno 2016, che oggi rappresenta la data propria di scadenza delle concessioni attribuite più di recente sulla base della cosiddetta legge Bersani.

relativamente alla logica delle scadenze, ai bandi di gara connessi e alla possibile partecipazione del mercato europeo a questo tipo di gara.

Se così non dovesse essere, credo che né con la separazione delle reti, così come dimostrato (già la gara non aveva avuto successo), né con altri provvedimenti, se non quelli di un sostegno diretto a un settore in crisi, si potrà risolvere il problema del montepremi e della raccolta delle scommesse.

parere non ostativo, ad eccezione dell'emendamento l-*ter*.0.6, sul quale il parere è non ostativo, a condizione che, nel comma 6, sia esclusa l'individuazione degli organi regionali competenti ad emanare il regolamento, dal momento che ciò viola l'autonomia organizzativa delle Regioni, come ha affermato la Corte costituzionale in una giurisprudenza ormai consolidata. Con l'occasione, la Commissione evidenzia l'anomalia degli emendamenti 1-*bis*.2 e 1-*bis.*3, i quali, al comma 6, prevedono l'abrogazione unilaterale di norme contenute in convenzioni dì concessione, per le quali è previsto il coinvolgimento di soggetti privati. Inoltre, l'emendamento 1-*bis*.17 interviene a modificare una fonte di rango secondario con una norma di rango primario, mentre gli emendamenti 1-*ter*.0.100 prevedono, per l'adozione di un regolamento ministeriale, il parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari».

sugli emendamenti 1-*bis*.17, 1-*bis*.20 e 1-*bis*.21. Esprime un parere di semplice contrarietà alle proposte 1-*bis*.15 e 1-*bis*.16. Il parere è non ostativo sulle restanti proposte».

l'importanza dell'impegno nei confronti della lotta al rischio di infiltrazioni criminali nell'ambito delle attività legate al fenomeno dei giochi. È un tema su cui dobbiamo tutti essere particolarmente vigili e sul quale già opera significativamente la Guardia di finanza. Ma l'attenzione deve essere assolutamente alta. in sostanza, che il Governo si impegni «a mettere in atto tutte le misure necessarie per scongiurare ogni pericolo di infiltrazione criminale», a dare a dare vita ad apposite commissioni di monitoraggio e di verifica sulle attività illecite, con il compito di riferire periodicamente alle Camere, e a lavorare in collaborazione con la Guardia di finanza, puntando anche a destinare una quota dei proventi derivanti dal contrasto a tali attività illegali al rafforzamento delle dotazioni organiche della Guardia di finanza. Sinceramente, non capisco come queste richieste non possano essere accolte. Una raccomandazione,

G103 siano accolti come raccomandazione.

come evidenziato nella replica, ad iniziative chiare da parte del Governo sul tema del contrasto all'attività criminale, e in particolar modo al gioco illecito,

Faccio presente al sottosegretario Giorgetti, che che dopo questa discussione mi vorrà un po' meno bene, ma questo fa parte dei ruoli, che ho estrapolato letteralmente una frase che era contenuta nella relazione della commissione Grandi, quindi non mi sono inventato solo preso una frase che dava delle indicazioni operative e credo che sarebbe giusto andare in quella direzione. Tuttavia, per il bene che voglio alla Guardia di finanza - e credo che questa sia una posizione che unifica il nostro Gruppo - accetto la riformulazione perché rimane il tema dell'impegno e del sostegno alla Guardia di finanza.

insiste per la votazione

per quanto riguarda l'UNIRE. È in corso una verifica dei conti circa le condizioni dell'UNIRE, il Governo chiaramente si riserva, compiuta questa verifica, di intervenire nel senso che è già indicato all'interno del decreto. Ritengo pertanto francamente che la votazione di quest'ordine del giorno sia una votazione del tutto inutile, perché già all'interno del testo si possono raccogliere gli elementi sulla volontà del Governo che va in tal senso.

Tutti gli emendamenti sopra richiamati di carattere aggiuntivo non attengono, infatti, all'attuazione di obblighi comunitari come, invece, previsto dal decreto-legge, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Sinceramente non si capisce perché la dilazione temporale sia stata così prolungata e rinviata fino alla scadenza del luglio del 2009. È vero che c'erano sette mesi di termine tecnico, ma essendo la gara stata assegnata nel marzo i sette mesi sono largamente superati. Tra l'altro, le motivazioni che risultano dalla relazione tecnica lasciano intendere che chi va vinto e si è aggiudicato la gara doveva mettere a punto una serie di nuovi requisiti. Resta quindi il dubbio se li aveva o no per poter vincere la gara, ma soprattutto rimane il tema

delimitare l'ambito di un'operazione che, secondo noi, davvero ha esorbitato rispetto alle prescrizioni che dovevano in qualche modo portarci a rientrare dall'infrazione comunitaria. Sono 329 le agenzie ippiche che devono essere superate. Si coglie l'occasione, con questa operazione, per compiere una riorganizzazione complessiva per 3.000 punti, andando ad una revisione delle convenzioni in essere. Si prefigurano altresì *benefit* - come diremo dopo - per chi è già titolare di una concessione e può quindi giovarsi di uno sconto per rientrare in questa nuova possibilità

di comportamenti non regolari, per combattere la diffusione del gioco illegale, l'evasione e l'elusione fiscale, oltre che per garantire la tutela del giocatore. Prima di concludere, vorrei mettere in evidenza un emendamento che sta particolarmente a cuore

una possibilità di vedere riassegnati i fondi che la specifica tabella collegata alla finanziaria ha fatto venir meno (circa 115 Il motivo credo sia molto condivisibile. So quanto il Governo e il Parlamento tengano allo sport italiano, all'attività delle federazioni sportive nazionali e delle strutture complessive del CONI. Confido quindi in un positivo accoglimento dell'emendamento

e per evitare che il decreto-legge decada.

Presidente, chiedo di aggiungere la mia firma a questo emendamento e anche di fare, eventualmente, una dichiarazione di voto.

il senatore Barelli ha illustrato l'emendamento, che il relatore si è rimesso al Governo e che quest'ultimo ha chiesto al presentatore di trasformarlo in ordine del giorno. Io chiedo di aggiungere la mia firma e di poterlo presentare a mio

del presidente del CONI Petrucci, che ha illustrato le condizioni del prossimo quadriennio olimpico del CONI in conseguenza del taglio di 112 milioni di euro in finanziaria.

una componente non irrilevante degenera nei suoi comportamenti e il gioco diventa una forma patologica,

per porre fine soprattutto a quelle forme degenerative del gioco, delle quali ci dobbiamo occupare dal punto di vista psicologico e psichiatrico.

gli interessi erariali in gioco, cercando in primo luogo di fare salva (questo il testo delle integrazioni che proponiamo all'articolo), nell'interesse dell'erario, la possibilità di svolgimento di attività di verifica delle connessioni in rete del parco macchine e di eventuali azioni di recupero

ne spiego le ragioni. Il Governo, ancora una volta, è stato sordo e cieco nel non accogliere alcuni emendamenti che potevano che potevano contribuire a battere quella che è la piaga della dipendenza. Basta leggere alcuni giornali

La psicologa del SERT: "Il pericolo da *videopoker* e cavalli". Al Lotto più si scommette, più si perde».

Lega Nord è sensibile a questi problemi. Lo voglio ripetere ancora oggi: c'è un grave allarme sociale un grave allarme sociale e lo Stato diventa una sorta di biscazziere, perché incamera ingenti risorse

La diffusione globale del gioco d'azzardo trova conferma nella stessa etimologia della parola "azzardo" che deriva dal francese "*hasard*", una parola a sua volta di origine araba derivante dal termine che designava il dado, uno dei più antichi oggetti a cui si lega la tradizione del gioco sociale di scommessa. Lo sviluppo sociale del problema del gioco d'azzardo è in parte favorito anche dalle crescenti possibilità di scelta tra una vasta gamma di tipologie di gioco, ormai sempre più legalizzate, che riescono a rispondere alle simpatie dei giocatori con diverse propensioni e con differenti personalità. Così, i giocatori d'azzardo vanno dagli amanti della trasgressione da gran salone, come quella dei giochi da casinò e delle *slot machine*, agli appassionati dei videogiochi, che si lasciano conquistare dai sempre più diffusi videopoker, agli appassionati dei giochi d'azzardo popolari, come le lotterie, il gioco di numeri e di schedine, fino al Bingo, la moderna trasformazione del gioco della tombola, che riesce a conquistare anche interi gruppi grazie al suo profondo legame con il vissuto di una concessa usanza festiva a dimensione familiare. Per chiarire le caratteristiche diagnostiche del gioco patologico - lo ha ricordato anche la senatrice Baio - è importante distinguere il vizio del gioco dalla malattia del gioco, sottolineando anche che spesso esiste una tendenza ad usare il primo termine per designare impropriamente comportamenti patologici. La distinzione è importante perché permette di individuare una delle caratteristiche fondamentali del gioco d'azzardo patologico (disturbo siglato in psichiatria), vale a dire la perdita di controllo sul proprio comportamento, che invece nel vizio è un comportamento volontario, che può essere controllato ed eventualmente interrotto da una persona che, tuttavia, lo mette in atto con volontà e consapevolezza delle connotazioni negative attribuite ad esso da un punto di vista morale. secondo i criteri classificatori tradizionali della psichiatria, possiamo sintetizzare che siamo in presenza di gioco d'azzardo patologico quando esiste un comportamento persistente, ricorrente e disadattivo di gioco d'azzardo, intendendo in quest'ultimo caso che il gioco è in grado di avere delle pesanti ricadute negative sulla vita personale, sociale e lavorativa del giocatore.

per appaltare l'istruzione pubblica ai privati, mentre trova fondi sufficienti per il decreto salvabanche per dare contributi agli istituti di credito ed ai lauti stipendi dei banchieri, non trova in alcun capitolo di spesa risorse per salvare le famiglie impoverite, che devono ricorrere al debito o all'illusione del gioco per sopravvivere. Anzi, con il decreto-legge n. oggi in discussione in Aula, il Governo incentiva lo Stato biscazziere, ritenendo che la soluzione dei problemi delle famiglie che soffrono una delle più gravi crisi economiche del dopoguerra, con la perdita dei risparmi e dei posti di lavoro,

giocatori ha una dipendenza dal gioco, fenomeno che si aggrava nelle fasi economiche di recessione e che investe soprattutto le fasce di popolazione più povere e con meno disponibilità finanziaria, come le donne, le casalinghe, i pensionati, con casi in cui si arriva a indebitarsi per alimentare il vizio del gioco e perfino a perdere la casa per pagare i debiti da gioco. Concludo, signora Presidente, onorevoli colleghi, affermando che questo Governo sbaglia ancora una volta ad approvare un decreto-legge che non prevede alcuna forma di tutela per i deboli e gli anziani e commette un tragico errore ad alimentare lo sfruttamento del vizio da parte di uno Stato biscazziere che avrebbe il dovere di salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie con strumenti più incisivi delle scommesse e delle lotterie.

definita e chiara. È un terreno difficile, sul quale in parte possiamo solo condividere quanto sostenuto poco fa dal collega Lannutti;

settori. In questo caso, lasciando perdere la parte più tecnica del decreto che andiamo a convertire quest'oggi (quindi quel richiamo ad adeguarsi a norme e ad inviti della Comunità europea affinché le procedure di gara avessero l'evidenza richiesta dalle norme europee),

lavoro si è fatta promotrice in prima persona la Lega Nord. Non si può fare di tutta l'erba un fascio, dicendo che i giochi e le scommesse sono in assoluto qualcosa di deleterio. Essi sono utili, come in questo caso, a sostenere un settore economico, sportivo, culturale sociale molto importante. Per questi motivi, e con la soddisfazione di rivendicare da parte del movimento politico cui appartengo e del ministro Zaia una grande attenzione al mondo dell'ippica e dell'allevamento dei cavalli e delle razze equine, confermo ovviamente il voto favorevole della Lega Nord.

lamentando come in Senato i tempi di esame di questo provvedimento siano stati ridottissimi, soprattutto per la Commissione di merito, che non ha potuto disporre dei pareri delle altre Commissioni, anche su aspetti di rilievo. Che i tempi siano stati ridotti lo dimostra anche il fatto che la stessa maggioranza, per trovare un'intesa, ha dovuto chiedere una sospensione dei lavori d'Aula.

Poiché parliamo di giochi, mi arrischio a scommettere, tanto per restare in tema, che di qui a breve saremo chiamati a correggere e precisare alcune delle disposizioni contenute nel provvedimento. Venendo al merito, vi sono alcune cose che non convincono. Ho già detto delle perplessità in ordine all'ampio spostamento in avanti della decorrenza della nuova concessione per la gestione da parte della SISAL dell'esercizio del gioco dell'Enalotto. Qui si fa davvero un regalo importante al nuovo soggetto gestore, non so se per trascuratezza

contro i poteri forti e di rastrellare qualche risorsa nell'interesse dell'erario. Invece, scopriamo che quando c'è da stringere al Ministero dell'economia l'*animus pugnandi* è più o meno quello di un don Abbondio e non va molto più in là di questo criterio e di questa regola. Anche per quanto riguarda il rispetto delle normative comunitarie, abbiamo già avuto modo di discuterne ma qui si è colta l'occasione di ovviare a un'infrazione comunitaria ampliando, però, in maniera talmente rilevante la riorganizzazione da disegnare un nuovo assetto del sistema. Non si è però prestata attenzione ad elaborare quelle valutazioni

orientare le scelte in funzione di individuare nuove modalità di distribuzione del gioco su base ippica allo scopo di combattere la diffusione di quello illegale, l'elusione e l'evasione fiscale oltre che garantire i giocatori.

aspetto: noi rischiamo, per evitare una sanzione della Comunità europea, di incorrere in un'altra infrazione. Non si giustifica diversamente, e non si comprende se non come un favore fatto a qualche altro interesse cui si vuole in qualche modo compiacere, lo sconto nei nei confronti di quei soggetti che, già titolari di concessione, se partecipano alla gara potranno abbattere il costo degli 85.000 euro del 25 per cento: è una regalia sinceramente, non si comprende il motivo. Ribadisco che si sarebbe dovuto esercitare un controllo molto più severo circa il fatto che questi soggetti abbiano ottemperato correttamente a quegli obblighi che l'essere titolari di convenzione riconosceva alla loro responsabilità.

Noi siamo favorevoli al fatto che si sia trovata la maniera di sostenere un settore in sofferenza, quale quello dell'allevamento dei cavalli. Da questo

Detto questo, ho l'impressione che nel definire la provvidenza si sia forse ricorsi a una misura *extra large*. Non so se qualcuno ha fatto bene i conti ma quel testo è scritto in una maniera certamente per iniziati e non per persone che possano agevolmente comprenderlo. Secondo me, esso contiene anche delle formulazioni che saranno fonte di ambiguità e di incertezza. Soprattutto, ritengo che non si siano fatti bene i conti. Io, allora, ho provato a rifarli:

se si stabilisce un aggio ulteriore dello 0,70 su quella base e se si presume che la base del gettito non diminuisca (bisogna infatti sapere che molte macchinette non sono collegate e non sono state portate a

così largheggiato nel dimensionamento di questo sostegno, che andrà ben oltre le previsioni e le intenzioni, e poi non si trovino da parte del Governo 20 milioni per garantire ai ciechi di guerra l'indennità sostitutiva dell'accompagnatore militare, si neghino le garanzie per il recupero dei crediti vantati dalle aziende italiane nei confronti dei Paesi stranieri, si taglino del 32 per cento le risorse del Fondo per le famiglie. Anche queste sono scelte politiche

che almeno a campione analizzino e sanzionino eventuali irregolarità. Vorremmo che, mentre si riprende - speriamo - una riflessione sulla riforma dell'Agenzia dei monopoli di Stato, che è stata prevista dalla finanziaria del 2008, si attivi fin da subito una specifica direzione di vertice incaricata di occuparsi di accertamento, discussione e contenzioso, un organismo centrale di *audit* che consenta di tenere sotto monitoraggio i comportamenti,

e alla tutela dei giocatori, all'introduzione di misure di contrasto e di sostegno contro le patologie di dipendenza, alla promozione di campagne di informazione e di sensibilizzazione volte a mettere in guardia contro le insidie dei giochi e le più sofisticate forme di cattura delle potenziali prede. Come si vede, signor Presidente, il Partito Democratico considera necessario un approccio molto più rigoroso e complessivo al tema, di cui non ci sfuggono la rilevanza ma anche i profili di criticità. Spiace dover constatare che anche in questo caso Governo e maggioranza abbiano preferito intervenire con misure approssimative, poco coordinate, tradendo la volontà di incentivare comunque il gioco e forse strizzando l'occhio a qualche interesse particolare. Questa è una responsabilità che vi lasciamo per intero.

mi coinvolge invece per la responsabilità che abbiamo noi tutti parlamentari di fare delle buone leggi. Il provvedimento al nostro esame è una buona legge se ci atteniamo allo scopo della legge stessa, che era quello di recare urgentemente delle disposizioni in modo da adempiere

nell'altro ramo del Parlamento per estraneità di materia, considerato comunque che bisognerebbe forse intervenire sul gioco, vi facciamo osservare che se il gioco è una droga, come dice il senatore Lannutti, allora bisognerebbe comportarsi

A questo punto, visto che non siamo d'accordo, se la tossicodipendenza bisogna affrontarla in modo diverso rispetto alla ludopatia, la ludopatia bisogna affrontarla così come stiamo facendo noi, cioè prevedendo un'irregimentazione delle disposizioni, con opere di manutenzione e cercando di cogliere un obiettivo che

sulle proposte che sono state fatte non è di secondo piano. C'è un'attenzione tale per cui prossimamente, dice il Governo,

350.000 cavalli ci sono 75.000 addetti, quindi circa 5.000 famiglie. E si tratta non solo di famiglie di scommettitori, ma anche di famiglie di autotrasportatori, di giardinieri, di sellai, di manutentori, di addetti alle ditte di abbigliamento. Con questo provvedimento, quindi, si sta operando un intervento di tipo socio-economico di non secondaria importanza. Si è, poi, cominciata a focalizzare la possibilità di introdurre, con un emendamento che poi è stato espunto nell'altro ramo del Parlamento, il gioco *on line*,

In ultimo, Presidente, con questo provvedimento andiamo verso la prevenzione delle tante distorsioni che ci sono nel settore e, quindi, il nostro scopo non è soltanto quello importantissimo di disporre una tutela del disporre una tutela del consumatore debole, ma anche quello, attraverso la lotta al gioco illegale, di garantire il gettito all'erario. Si compie una doppia azione che si configura

su una circostanza che il Gruppo del Partito Democratico considera alquanto grave. È in discussione, come lei e i colleghi sanno, presso l'8a Commissione del Senato,

In quella sede, il senatore Zanetta ha presentato un emendamento all'articolo 2 con il quale viene costituita la società Difesa Servizi Spa. Analogo tentativo era stato fatto presso la Camera dei deputati; il presidente Fini, in quella circostanza, ritenne di non dover ammettere la presentazione dell'emendamento per estraneità di materia. Ora, non che si debba pedissequamente emulare ciò che viene fatto nell'altra Camera, ma, a nostro giudizio, analogo atteggiamento dovrebbe tenere questa Presidenza, tenuto conto del fatto che, su un argomento che tratta di materiali e di contenimento dei prezzi, si vorrebbe in maniera surrettizia determinare una decisione del Senato che inciderebbe in maniera diretta e completa su tutta l'organizzazione della Difesa. Questo, dal punto di vista del merito; dal punto di vista del metodo, invece, signor Presidente, tutto questo avverrebbe senza che le competenti Commissioni avessero la possibilità di operare la seppur minima valutazione.

La seconda considerazione che vorrei fare è che, in prima istanza, ritengo che il giudizio sull'ammissibilità dell'emendamento debba essere espresso, a livello di Commissione, dal Presidente della stessa. Su questa base, poi, quando il testo arriverà in Aula, in sede di esame degli emendamenti, la Presidenza potrà esprimersi, altrimenti vi sarebbe un precedente pesante rispetto all'autonomia e al modo di lavorare delle Commissioni. Questi due aspetti mi pare si debbano entrambi tener presenti, quindi così ci comporteremo.

ho avuto modo di ascoltare uno dei pochissimi interventi degli esponenti di maggioranza in merito al disegno di legge sulla

più dopo la vittoria elettorale, il popolo italiano avrebbe chiesto con trepidazione ed urgenza di intervenire nel settore dell'ordine pubblico, perché la situazione d'insicurezza e di paura

soddisfacendo le legittime attese e pretese degli italiani. Penso che questo sia uno strano e furbo modo di porre la questione, innanzi tutto, come se la vittoria di una campagna elettorale legittimasse la maggioranza a fare di tutto, anche qualcosa che non corrisponde alle reali esigenze del Paese. Intanto, non abbiamo mai messo in dubbio la necessità che lo Stato sia sempre più presente, anche nel dare ai cittadini sicurezza e protezione. Ciò che ci divide dalla maggioranza, in questo momento, anche in questo settore, è il metodo che intende seguire, è la cultura che sottende a gran parte dei provvedimenti adottati, è il metodo scelto per assolvere a questo compito. Non ci siamo mai opposti in maniera pregiudizievole alla trattazione dei vari decreti e dei testi di legge; non l'abbiamo mai fatto in modo ideologico, rispetto a quelli che sin dall'inizio della legislatura voi della maggioranza avete imposto e state imponendo all'esame della Commissione, quindi dell'Aula, senza una riflessione ed un confronto approfondito. Quello che contestiamo è l'utilità e l'efficacia di buona parte dei provvedimenti che vi accingete ancora una volta a varare, forti solo della preponderanza numerica, senza confronto e riflessione, né una reale intenzione di affrontare il fenomeno sicurezza con serietà ed efficacia. Per ragioni di tempo formulerò alcune brevi riflessioni su alcuni degli istituti che intendete introdurre, anche perché il testo al nostro esame si presenta quanto mai eterogeneo, interessandosi di circolazione stradale, di norme sull'immigrazione, disposizioni sul contrasto al crimine organizzato ed intervenendo altresì sul cosiddetto regime speciale del carcere, previsto dall'articolo 41-*bis*, per gli appartenenti alle organizzazioni criminali di tipo mafioso. Si tratta di una sorta di zibaldone troppo variegato per essere particolarmente efficace. L'articolo 46 prevede il «Concorso delle associazioni volontarie al presidio del territorio». Nell'ipotesi normativa si prevede un'inutile possibilità che associazioni di volontari possano segnalare all'autorità di polizia eventi pericolosi per la sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale. Sottolineo che tale previsione è assolutamente inutile perché non è inibito ad alcuno segnalare o denunciare fatti e circostanze ritenute pericolose o situazioni di disagio sociale. Non vedo la ragione, al di là di una deprecabile azione politica di mera propaganda, per inserire in una norma ciò che che già possibile e legittimo fare da parte di singoli o di associazioni. La seconda parte della norma in esame prevede invece qualcosa di assolutamente illegittimo e pericoloso: l'istituzionalizzazione delle cosiddette ronde, gruppi di cittadini chiamati formalmente da parte degli enti locali (territoriali o no? A questa domanda sarebbe opportuno che il Governo fornisse una risposta chiara e immediata) a cooperare nello svolgimento dell'attività di presidio del territorio. Il provvedimento, se varato, sarebbe, come è stato in precedenza illustrato da altri colleghi del mio partito, contrario al dettato costituzionale, perché è demandato per legge alla competenza esclusiva delle forze dell'ordine il presidio del territorio, e sarebbe altresì pericoloso, proprio per la stessa sicurezza e per l'ordine pubblico. Il presidio del territorio, colleghi della maggioranza, è un compito così delicato e serio che in alcuni casi si è deciso, anche di recente,

requisiti che talvolta addirittura mancano persino nelle forze dell'ordine: so che sono casi eccezionali, ma è difficile avere serietà e professionalità da parte di chi è demandato a controllare il territorio. L'impiego in tale settore di ronde private, oltre ad essere certamente illegittimo si profila pericoloso, in quanto porrebbe un problema di *status* di compiti e di poteri delle persone impiegate e degli effetti che i loro atti produrrebbero anche nei confronti di terzi. Si richiama, a sostegno dell'istituto che si vuole varare, un altro istituto già noto da tempo al nostro codice penale, ossia l'arresto in flagrante di reato ad opera di privati, dimenticando l'eccezionalità di un simile istituto, che resta nella sua validità per ipotesi isolate ed eccezionali, in cui il privato che dovesse essere vittima o testimone di un reato grave o gravissimo possa trattenere il presunto autore del delitto per il tempo strettamente necessario a far intervenire la forza pubblica. Appare Appare del tutto anomalo ed errato servirsi e utilizzare la forza privata di un numero indefinito di associazioni come strumento stabile di collaborazione con compiti e poteri che resterebbero affidati solo alla fantasia di sindaci sceriffi o alla volontà di farsi giustizia da sé. Non stona rammentare, ad esempio, che proprio in questi giorni alcuni colleghi hanno presentato un'importante interrogazione sul modo in cui il Comune di Milano sta assegnando incarichi ad associazioni proprio in questo serio e delicato settore del presidio del territorio. In un momento in cui si profila peraltro la possibilità, anch'essa imposta dalla maggioranza, di reintrodurre il delitto di oltraggio al pubblico ufficiale, non si può fare a meno di chiederci chi sono questi collaboratori per il presidio del territorio e come verranno strutturati, inquadrati ed organizzati. Quale sarà il loro *status* giuridico? Saranno esercenti di un'attività di pubblico interesse o addirittura pubblici ufficiali? con quali conseguenze in un momento in cui verranno a contatto con altri cittadini, reali o presunti autori di reato, verso i quali potranno usare anche la forza? forza? Entro quali limiti? Tutto questo non è detto nel disegno di legge. Penso che il problema dell'ordine e della sicurezza pubblica e, quindi, del contrasto ad ogni forma di illegalità sia un fatto tanto serio da non consentire, amici della maggioranza, interventi errati e pericolosi come questo che state proponendo. Nel testo di legge in esame si reitera ancora una volta la cultura della repressione, tutta e solo basata sull'uso della forza, la repressione fisica, intesa non come l'*extrema* *ratio* di una necessità assoluta ed urgente di rispondere ad atti aggressivi e pericolosi non altrimenti neutralizzabili, ma come terapia sempre più Lo stesso criterio viene seguito nei confronti del fenomeno migratorio, quanto mai complesso, alla cui base vi sono atti di ingiustizia e di violenza, alcuni dei quali, giova ricordarlo in questa sede, si sono sedimentati nell'arco di secoli a danno di intere popolazioni e continenti,

che si pone talvolta come la conseguenza storica di errori e violenze perpetrate dai popoli privilegiati a danno dei più sfruttati e poveri. Eppure, a fronte di tale fenomeno, l'attuale maggioranza non sa offrire altra risposta al di fuori di una sterile ed inutile politica della repressione. Prima si inventa un delitto di immigrazione clandestina che, se varato, avrebbe imposto la celebrazione di decine di migliaia di processi e relative incarcerazioni, con conseguente ulteriore paralisi del sistema già compromesso della nostra giustizia. Ora si tira fuori una contravvenzione penale, che comunque imporrebbe l'esercizio dell'azione penale, da ritenersi estinta o interrotta solo nell'ipotesi di eseguita espulsione. Quando passeremo all'esame degli emendamenti approfondiremo questo aspetto e vedremo di che natura è l'intervento punitivo o l'oblazione, o la non oblazione, di questa contravvenzione. Anche in tal modo appare tutta l'approssimazione e l'inutilità dei sistemi prospettati nel disegno di legge; strumenti inutili e dannosi per gli effetti devastanti sul già provato e quasi paralizzato sistema giudiziario; decine di migliaia - tanti sono - di processi da attivare dinanzi ai giudici di pace con una duplice, inutile conclusione: o il processo si concluderà, con quali tempi non è possibile prevedere, ovvero interverrà l'espulsione, con la conseguente estinzione delle procedure. E se di estinzione si potrà tecnicamente parlare, In entrambi i casi, chiedo ai colleghi della maggioranza quale sarebbe il risultato, quale sarebbe il vantaggio per la nostra società. Trattandosi di una moltitudine di disperati, il più delle volte in possesso solo di laceri indumenti, quali possibilità in realtà, che paghino l'ammenda? Ma se non pagassero si dovrebbe procedere alla conversione della pena pecuniaria in detentiva! E se invece il soggetto verrà realmente espulso, quale necessità vi è stata di ingolfare le aule di giustizia, già fin troppo congestionate, con un mare di inutili procedure? Sin dal primo decreto sulla sicurezza che avete varato, abbiamo tentato, inutilmente, di contribuire ad una più utile e corretta impostazione delle norme proposte, consigliando l'introduzione, ad esempio, dell'istituto del rimpatrio assistito, assistito, che nel nostro Paese ha già trovato una proficua attuazione al tempo della guerra del Kosovo. L'attuazione di un simile istituto varrebbe certamente ad evitare abusi e vessazioni verso chi di violenze e di ingiustizie ne ha già subite troppe e anche ad utilizzare le risorse pubbliche con maggiore parsimonia e proficuità. Ricordo infatti che il trattenimento nei centri di identificazione e di espulsione costa più del sostegno per un rimpatrio assistito. Il persistente diniego della maggioranza non trova alcuna giustificazione se non la pervicace, sterile volontà di mostrare i muscoli anche quando appare chiaramente come lo strumento meno idoneo a risolvere il problema. La politica dei muscoli, della cosiddetta tolleranza zero, riappare ancora una volta, dopo l'esperienza dei campi rom, anche - sembra impossibile crederlo - nei riguardi dei senza fissa dimora. Si tratta di una categoria di cittadini, di persone tra le più povere e certamente escluse dai più elementari servizi essenziali che la società moderna offre, persone che vivono per strada, che portano con sé tutto il loro misero patrimonio. Nei confronti di tale persone, certamente sfortunate e deboli, sarebbe stato auspicabile ed apprezzabile un'iniziativa del Governo diretta alla conoscenza del fenomeno per definirne le cause e l'entità dello stesso, cercando i possibili rimedi. Nulla di tutto ciò, perché il «Governo forte» di centrodestra, quello che dice di farsi rispettare e di tolleranza zero, decide dare vita ad un registro in cui tutti i pericolosi *clochard* - i barboni - dovrebbero essere inseriti: un registro da tenere presso il Ministero dell'interno e non degli interventi sociali, una vera e propria schedatura che non si comprende a quale fine, con quali risultati e per la sicurezza di chi! Non risulta infatti - almeno le cronache non lo hanno mai evidenziato - che uno o più persone di questa categoria si siano resi responsabili di crimini o reati di ogni genere. Quindi, continuiamo a chiederci la ragione di un simile atteggiamento repressivo anche quando non serve o addirittura si concretizza con provvedimenti disumani. Non piani di sostegno ma interventi repressivi. Ed ancora un'ultima perla. Secondo la stessa concezione, si prevede il *test* di lingua italiana come condizione per il rilascio del permesso di soggiorno di lunga durata: ad una moltitudine di disperati, assai spesso privi di una cultura di base anche del loro Paese e nella loro lingua, imponiamo, come requisito necessario per ottenere il permesso di soggiorno a lunga scadenza, la conoscenza della lingua italiana; e non pensiamo invece ad organizzare sistemi che favoriscano l'apprendimento della lingua, ma non

Siamo aperti ad una collaborazione vera, siamo disponibili a fornire tutto il nostro sostengo per interventi, per istituti che servano all'obiettivo di regolare in maniera civile il processo di immigrazione, di di impedire o contenere le violazioni di legge, soprattutto quelle dei criminali, ma con istituti che non tocchino la dignità dell'uomo, che non facciano ridere l'intera Europa. questo che chiediamo. Quindi, almeno in Aula, apritevi alla riflessione, al confronto e al contributo attivo che siamo ancora disposti a fornire.

partirò dall'intervento del collega Maritati per chiedergli fondamentalmente in quale Paese surreale vive e quale Paese surreale ci sta dipingendo. Credo che sia finita l'epoca di pensare ad una immigrazione controllata e controllabile e che non vi sia davvero un'emergenza legata all'immigrazione clandestina. Il discorso delle ronde a cui il collega alludeva prima non nasce da una volontà della Lega scollegata dalla realtà, ma da una precisa esigenza il territorio. È il Paese che ci chiede e ci urla un bisogno di sicurezza, di sicurezza, che non è più garantita nelle nostre strade ma nemmeno nelle nostre case. Questo è quanto ci viene chiesto e questo è quello che abbiamo tentato di fare con l'emendamento sulle ronde e con tanti altri, atti a limitare l'ingresso incontrollato ed incontrollabile di una immigrazione che ci sta veramente mettendo in ginocchio, soprattutto dal punto di vista della sicurezza, perché l'immigrazione incontrollata e incontrollabile, alla fine,

Questo è il significato di tutta una serie di emendamenti che abbiamo voluto fortemente portare avanti per potenziare in senso ancora più restrittivo

Un altro nodo dibattuto in Commissione ma anche sulla stampa è quello del permesso a punti e ancora di più lo è quello dell'obbligo di denuncia nei pronto soccorso dei cittadini extracomunitari clandestini, conseguente all'introduzione del reato di clandestinità, che ritengo assolutamente sacrosanto. E non è dimostrazione di razzismo o di menefreghismo nei confronti del cittadino sofferente il fatto di andarlo a denunciare: sono due cose distinte e separate. Un conto è il diritto alla salute, che non viene negato assolutamente a nessuno: nei nostri pronto soccorso tutti i cittadini, siano essi italiani o extracomunitari, ricevono le cure più premurose e le migliori possibili in quel momento, le vite umane vengono salvaguardate, le malattie vengono curate; ma se quello della salvaguardia della salute è un diritto, è altrettanto un diritto da parte nostra, dei cittadini di questo Paese, che la legalità venga comunque rispettata. La clandestinità è di per sé aberrante;

venga a conoscenza dell'esistenza di un reato ha l'obbligo morale, civile e civico di segnalarlo all'autorità giudiziaria perché vengano presi vengano presi tutti i provvedimenti necessari per provvedere ad una rapida e duratura espulsione dal nostro Paese di individui che evidentemente sono qui solo ed esclusivamente per compiere reati. Volevo solo puntualizzare questo piccolo particolare per fugare ogni dubbio e separare, una volta per tutte, la necessità di venire incontro ad un bisogno sanitario, dalla necessità, sacrosanta e sancita, di venire incontro al bisogno di sicurezza e alla limitazione di questa immigrazione, che ormai sta diventando selvaggia. Siamo alla resa dei conti: o riusciamo a fermarla adesso o non avremo una seconda occasione.

perché, come abbiamo sentito dal collega, la clandestinità è delinquenza. Quindi, tutte le badanti che sono nelle nostre case, tutti i muratori che lavorano nei nostri cantieri ed i pizzaioli, che sappiamo essere clandestini perché con la Fini-Bossi sono anni che non riescono a regolarizzarsi, sono delinquenti. Sono 700.000, caro collega: lei pensa di fare 700.000 accompagnamenti forzati o di metterli in carcere? Perché il punto di tutto il ragionamento che abbiamo fatto fino adesso è questo:

questi temi cercando di nascondere sotto il tappeto il problema dei problemi: la Fini-Bossi è fallita. Non c'è problema, posso anche dire che la Turco-Napolitano è fallita, dal punto di vista del tentativo di definire quote e blocchi di ingresso e di regolare. Dobbiamo allora sederci intorno ad un tavolo; se c'è un problema *bipartisan* dovrebbe essere questo, perché è il problema del nostro futuro e del futuro dell'Europa. È un problema che riguarda tutte le società Possiamo far finta di affrontarlo come se ci fosse capitato un accidente a cui cerchiamo di porre mano? Siamo già ai bimbi della seconda generazione, siamo già ai matrimoni misti, ad un'evoluzione della popolazione; dobbiamo affrontare questa tematica guardandola in faccia, per quella che è, cercando di evitare l'immigrazione non regolata ma dando il massimo di opportunità di integrazione e di cittadinanza a chi è qui per lavorare. Vede, le sue parole, senatore Rizzi, ci fanno capire quanto siano mi perdoni - poco sincere tutte le espressioni, non sue, ma di molti suoi colleghi, che quando sentono le nostre critiche ci dicono: «Per chi viene qui a lavorare onestamente, braccia aperte; in galera». E tutti dicono: «Giusto, i delinquenti devono andare in galera e se sono stranieri devono essere espulsi e tornare Ma poi sentiamo dalle sue parole e leggiamo dai testi di legge che vengono qui proposti che non sono solo i delinquenti: tutti tutti coloro che sono clandestini sono potenzialmente delinquenti. Questo è un errore culturale molto grave, perché ogni volta che viene avviata un'indagine o un'inchiesta lei scoprirà che tanti delinquenti stranieri - lasciamo perdere gli italiani, in questo momento - hanno tanto di permesso di soggiorno e di timbri

merito ad un bando sul controllo del territorio emesso dal Comune di Milano. Ho l'onore di venire da una città che anticipa molto. molto. Questo bando per il controllo del territorio in collaborazione con le forze dell'ordine è stato vinto da due associazioni:

l'altra è un'associazione di ex poliziotti il cui presidente è un nostro collega consigliere comunale di Forza Italia. Al di là

ho provato a rileggere tutti gli articoli che parlano degli stranieri e non quelli che parlano di delinquenza, anche se ci sono fenomeni di delinquenza connessi all'immigrazione, come sempre quando ci sono grandi movimenti migratori (e noi italiani ne sappiamo qualcosa); in questo testo di legge ci sono quindi articoli sacrosanti che centrano problematiche riguardanti reati connessi alla tratta e a tutti i fenomeni che, purtroppo, in molte situazioni accompagnano i grandi fenomeni migratori. Mi riferisco però agli altri, a quelli che non c'entrano niente.

Perché le condizioni igienico-sanitarie necessarie per avere l'iscrizione anagrafica devono trovare collocazione in un provvedimento sulla sicurezza? Perché l'opportunità che gli stranieri imparino la lingua italiana, eccetera,

che si sta cominciando a delineare una specie di doppio diritto. Sono molto fiera di vivere nel mondo occidentale e semmai dovessi poter vantare degli elementi di superiorità culturale

di doppio diritto, dove ci sono delle persone che, pur vivendo qui regolarmente, rischiano di perdere i diritti da un momento all'altro?

di cui, piaccia o non piaccia, il nuovo Presidente degli Stati Uniti è lampante protagonista e che è un futuro a cui dobbiamo guardare. Possiamo anche pensare di chiuderci in casa,

larghi strati di popolazione possono aver paura ad affrontare questo futuro. Ma il compito di una classe dirigente è accompagnare verso il futuro,

Mi viene in mente - tanto siamo qui praticamente tra amici, per cui possiamo anche lasciarci andare - l'antica Sparta. Io non voglio vivere in una società che assomiglia a Sparta, con gli spartiati che hanno tutti i diritti, gli iloti liberi, ma senza diritti civili, e una moltitudine di schiavi.

con un appello, se possibile. Signor Sottosegretario, Governo, amici della maggioranza, svolgere una sessione sulla situazione dell'immigrazione in Italia e in Europa, con i dati alla mano, vedendo quali sono i fenomeni? Al collega

Vogliamo confrontarci con questi fenomeni? Vogliamo decidere che a quelli che lavorano qui, che hanno il permesso di soggiorno, che hanno tutti i santi crismi e sono onesti concederemo la cittadinanza e il diritto di voto, favorendo i ricongiungimenti? O pensiamo di spingere anche loro in una sorta di precarietà? Io ho letto un signore che si chiamava Carlo Marx (lo abbiamo letto in pochi), quale parlava di esercito di riserva. Dobbiamo ritrovarci lì? Con dei lavoratori in una fascia grigia che teniamo come esercito di riserva e che hanno dei diritti solo se noi siamo così ricchi da non aver bisogno, ma che siamo pronti a buttare a mare

mi preme innanzitutto esprimere il mio consenso e il mio appoggio all'impianto generale del disegno di legge all'esame, che forse per la prima volta, in maniera adeguata e secondo le necessità, offre strumenti necessari per garantire ai cittadini tranquillità, serenità e la possibilità

i senatori Coronella, Sarro, Vetrella, Compagna, Sibilia, Esposito, Izzo e Calabrò. Si tratta dell'emendamento 48.0.107, che sostanzialmente riassume un mio vecchio disegno di legge, che approdò anche all'Aula due legislature fa e che ho riassunto sotto forma di emendamento perché fosse esaminato in questo contesto. Chiedo perciò all'Assemblea e, in modo particolare, al rappresentante del Governo di dedicare a questo emendamento una particolare attenzione, perché credo che, se approvato, signori relatori, possa rappresentare uno strumento agevole, di trascurabile impegno finanziario, ma di straordinaria efficacia nella lotta alla criminalità organizzata. Voi tutti avrete sicuramente seguito le vicende relative all'ultima, recente strage di camorra avvenuta sul litorale domizio, nel Comune di Castel Volturno, e le drastiche misure che sono state immediatamente adottate per fronteggiare in maniera efficace, nell'area della Provincia di Caserta, la tragica, sanguinosa, crudele ed inammissibile avanzata della criminalità organizzata. In quel territorio, onorevoli colleghi, come saprete, lo Stato e le stesse istituzioni democratiche sono quotidianamente aggredite e spesso calpestate ed umiliate da *clan* camorristici, tra i quali tristemente primeggia, per ferocia, capacità e forza intimidatorie, quello tristemente noto come *clan* dei Casalesi. La Direzione distrettuale antimafia, la Direzione da tempo sono impegnati per combattere quelle forze del male e non di rado riescono ad ottenere, con grandi sacrifici e con encomiabile impegno, risultati a volte insperati. Tutto ciò però non è ancora sufficiente, perché la criminalità camorristica è tuttora forte, pressante ed incombente su una popolazione che avverte questa presenza e che spesso, impotente ed impaurita, rimane annichilita, soffrendo l'angoscia quotidiana di rimanere vittima di atti di violenza e di sopraffazione. Le ultime, recenti misure hanno sicuramente stretto la morsa intorno alla vasta area delinquenziale, tant'è che hanno portato all'arresto di molti latitanti e alla individuazione dei responsabili di numerose gesta criminali. Ma non basta, perché la straordinarietà dell'intervento è purtroppo destinata ad essere limitata nel tempo, anche se ci auguriamo che le forze dell'ordine lascino quel territorio dopo che avranno ristabilito in maniera accettabile e duratura la legalità. Bisogna allora pensare anche a riforme strutturali che migliorino il sistema e lo rafforzino. Bisogna pensare, in particolare, ad un sistema giudiziario con una consistente e significativa presenza territoriale, che riesca ad intervenire ed a mettersi in moto in tempi rapidi, dando risposte pronte ed eliminando allo stesso tempo sprechi di risorse umane e finanziarie, oltre a difficoltà strutturali ed organizzative. Onorevoli colleghi, attualmente i reati di matrice camorristica sono di competenza della Direzione distrettuale antimafia di Napoli che ha giurisdizione su tutto il distretto della corte di appello di Napoli, su una popolazione cioè che comprende le Province di Napoli, Caserta, Salerno, Benevento ed Avellino: vale a dire circa 5 milioni di abitanti. Una corte che ha quindi dimensioni mastodontiche, di gran lunga superiore all'*optimum* generalmente indicato dagli esperti di organizzazione giudiziaria. A ciò si aggiunga, ai fini della condivisibilità e sostenibilità dell'emendamento 48.0.107 (per la cui approvazione io mi rivolgo a tutta l'Aula, indipendentemente dalle barriere o barricate politiche che possono essere alzate), che ben il 40 per cento dei reati di camorra, signor rappresentante del Governo, vengono purtroppo consumati sul territorio casertano e che una pari percentuale di imputati vive e delinque in Provincia di Caserta. Attualmente, pertanto, tra l'altro, accade che magistrati della Direzione distrettuale antimafia di Napoli istruiscono processi per i quali, al momento del dibattimento, quasi sempre, in maniera sistematica, direi, vengono poi delegati, per sostenere l'accusa, magistrati del tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Il che significa che il magistrato delegato, quello appunto di Santa Maria Capua Vetere, oltre ad essere sottratto al suo non lieve lavoro ordinario, deve leggere e studiare gli atti, sempre ponderosi, complessi e impegnativi, che già aveva formato, letto e studiato il suo collega della Direzione distrettuale antimafia: insomma, una inutile, faticosa e dispendiosa reiterazione che appesantisce ancora di più quella elefantiaca e lentissima macchina che è diventata la giustizia. E ciò senza considerare che non di rado i magistrati della procura di Santa Maria Capua Vetere vengono delegati anche per attività di indagini, specie per quelle relative a processi di competenza della Direzione distrettuale antimafia ma iniziati o promossi dai pubblici Con l'emendamento 48.0.107 in discussione si costituisce una nuova corte di appello in Caserta (che - faccio notare - è l'unico capoluogo di Provincia a non essere sede di tribunale: un fatto unico che si perpetua ormai nei decenni), e quindi, tra gli altri uffici che accompagnano questa istituenda corte di appello, vi sarebbe anche una Direzione distrettuale antimafia, con giurisdizione sui tribunali di Santa Maria Capua Vetere, Ariano Irpino e Nola, vale a dire su una popolazione di un milione di abitanti, che è un numero di persone che potremmo definire un ufficio di dimensioni ottimali, rispetto alla effettiva domanda di giustizia di quella comunità, tenuto conto delle condizioni socio-economiche, del flusso dei procedimenti, del tasso di criminalità comune ed organizzata e, soprattutto, di alcune peculiarità locali che, ritenute straordinarie fino a pochi anni or sono (tant'è che per molti anni si è parlato di "fenomeno" della criminalità organizzata, a sottolineare la sua specificità, la sua straordinarietà), sono purtroppo diventate ordinarie. La istituzione della nuova corte di appello, inoltre, rafforzerebbe, proprio in maniera fisica, la presenza dello Stato e rappresenterebbe un altro visibile e prestigioso simbolo della legalità. Le popolazioni interessate e gli operatori del settore, signor rappresentante del Governo e signori relatori, ora stanno seguendo con viva apprensione questo momento ed attendono con straordinaria ed encomiabile fiducia che il Parlamento non li trascuri, anzi li aiuti a continuare a credere nello Stato, nella legalità e a coltivar l'ormai arida pianta della speranza. Onorevoli senatori, da casertano e soprattutto da chi in quell'area ha operato come magistrato per moltissimi anni e sempre in territori difficili, sono fermamente convinto e vi assicuro che l'innovazione che caldeggio e che insieme a me sostengono anche i senatori che prima ho nominato (che fra l'altro alleggerirà in maniera consistente l'enorme mole di lavoro della corte di appello di Napoli) rappresenti uno strumento particolarmente duttile ed efficace per fronteggiare e combattere la criminalità organizzata. Questa mia ferma convinzione, unitamente ai voti di una popolazione che attende con fiducia che lo Stato mostri il suo interesse e la sua partecipazione verso la straordinarietà di una situazione divenuta angosciante, mi induce a chiedervi in maniera veramente accorata il sostegno di tutti. pertanto tutti i colleghi a guardare con attenzione a questo caso. È un momento forse unico per la Provincia di Caserta perché possa essere offerto a quel territorio uno strumento

dieci *flash* le preoccupazioni su questo provvedimento. Il collega Rizzi della Lega diceva prima che c'è una domanda sociale prorompente in termini di sicurezza. Nessuno nega che ci siano giustamente preoccupazioni di tenuta sociale, rispetto a questo tema, e paure da far scomparire con un'azione credibile dei pubblici poteri, però c'è modo e modo di farlo: non ogni modo può essere giustificato, in particolare non ogni modo corrisponde con gli intenti e con i valori della Costituzione, con i fondamenti culturali della nostra civiltà. con ordine. Ci sono cinque profili che ledono pesantemente le caratteristiche di dignità umana delle persone, tutelate nel nostro ordinamento. di legge, che subordina il rilascio di tutti gli atti di stato civile (compresi quelli relativi alla filiazione, ma anche al matrimonio) alla titolarità del permesso di soggiorno, pone limiti fortissimi alla tutela dei diritti civili primari lede, come ho già ricordato l'altro giorno, quel particolare primato della famiglia fondata sul matrimonio, che l'articolo 29 della Costituzione configura a difesa di forme troppo forti di invadenza dello Stato. È un punto chiave rispetto a questa normativa. In secondo luogo, l'articolo 47 del provvedimento, sul rimpatrio dei minori comunitari che esercitano la prostituzione, è irragionevole dal punto di vista della logica della norma,

che prevede misure del genere «soltanto in circostanze eccezionali, qualora vi siano motivi imperativi di pubblica sicurezza», come recita la direttiva, e quindi stiamo andando ad una violazione mediata dell'articolo 117 costituzionalità. Il terzo aspetto è quello del permesso di soggiorno a punti dell'articolo 41, il cosiddetto «accordo di integrazione» tra lo straniero e lo Stato: si rinvia il tutto ad un regolamento governativo per queste misure e ciò comporta una palese violazione dell'articolo 10 della Costituzione, che sancisce una riserva di legge, peraltro rinforzata, in materia di disciplina della condizione giuridica dello straniero. Per di più, non si escludono dalla possibilità di espulsione i titolari di protezione umanitaria, i rifugiati e gli asilanti, in chiara violazione del diritto internazionale e del diritto comunitario. Il quarto aspetto, il trattenimento dello straniero nei centri di identificazione e di espulsione (articolo 39, comma 1, lettera *l*) viola palesemente la direttiva della Comunità europea «*Migration Policy*», che invece si invoca a sostegno, la quale prevede che il termine massimo di diciotto mesi valga solo per i casi di resistenza all'identificazione, non per la mera difficoltà dell'accertamento. Inoltre, quinto ed ultimo rispetto a come il testo viola il principio della dignità umana, l'articolo 44 sulla schedatura dei *clochard* pone dei problemi molto seri, perché si rinvia tutto ad un mero decreto ministeriale, quando invece qui si tratta di dignità della persona e anche di tutela del dritto alla *privacy*. sono altri due aspetti nel testo vigente che violano invece la credibilità delle istituzioni. Vorrei insistere in particolar modo sulla questione delle cosiddette ronde di cui all'articolo 46, su cui anche oggi il periodico «Famiglia Cristiana» ha insistito in particolare per criticare questa legge, perché, vedete, quando noi creiamo un sistema in cui teorizziamo che, in nome del principio di sussidiarietà, delle realtà private entrino così in contatto sulla funzione di ordine pubblico e sicurezza, andiamo a colpire la credibilità di una risposta dello Stato e la logica stessa dello Stato, cioè il monopolio il monopolio legittimo dell'uso della forza. Con questo articolo è come se lo Stato si volesse spossessare di questo primato legittimo dell'uso della forza e ricorresse ad attività di privati per il presidio del territorio, in violazione dell'articolo 13 della Costituzione, che sancisce una riserva di legge rispetto all'adozione di provvedimenti limitativi della libertà personale che potrebbero derivare da questo concerto; e, per di più, qui c'è il problema dei limiti alla libertà di associazione e al divieto di associazioni paramilitari che viene in luce. L'altro aspetto (settimo punto), il secondo che va a colpire la credibilità dello Stato, è la norma-manifesto sull'immigrazione irregolare, che passa da reato penale, com'era nella prima versione, a reato amministrativo, ma in sostanza aggraverà il contenzioso giudiziario con l'unico effetto, uguale ad oggi, che ne conseguirà il provvedimento amministrativo dell'espulsione.

prevede, rispetto alle prestazioni sanitarie, che in caso di rifiuto del richiedente alla corresponsione di quanto dovuto, le strutture sanitarie ne trasmettano segnalazione all'autorità competente, quindi praticamente vincola il diritto alle condizioni economiche e fa una norma-fotografia della condizione di povertà, fondamentalmente di extracomunitari, per spingerli a non usufruire del diritto alla salute, nel timore di possibili conseguenze rispetto alle segnalazioni all'autorità competente. C'erano state versioni ancora più preoccupanti, rispetto al diritto all'assistenza sanitaria, ma questa resta profondamente incostituzionale e, direi, antiumana.

la cosiddetta disciplina dell'accordo di integrazione, che poi è il permesso di soggiorno a punti, anche agli stranieri che sono già in possesso del permesso di soggiorno e quindi con una *deminutio* dei loro diritti. Qui si incorre nel noto principio, rispetto alla tutela dei diritti civili e sociali, del divieto di *reformatio in peius*, cioè una volta conseguito un determinato standard di godimento dei vari diritti non si può recedere da questo livello, pena una profonda violazione del senso profondo della nostra Costituzione.

la locuzione «ben riconoscibili» rispetto a cittadini che magari non conoscono bene la lingua e che avranno difficoltà a difendersi dall'accusa di non essere ben riconoscibili? In conclusione, vorrei dire questo: i colleghi della Lega da cui derivano parte di queste iniziative hanno insistito, quando abbiamo esaminato il Trattato di Lisbona, con vari ordini del giorno sulle radici cristiane dell'Unione europea. Ora, sul termine radici cristiane si possono dire molte cose, dubito però che si possa parlare delle radici cristiane dell'Europa prescindendo dai criteri del giudizio finale di di cui al capitolo 25 del Vangelo di Matteo. Com'è noto, nei criteri del giudizio finale descritti nel capitolo 25 del Vangelo di Matteo si dice: «Ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere; ero forestiero e mi avete ospitato». A me non sembra che questa logica dell'«ero forestiero e mi avete ospitato» stia in varie parti di questo testo e, in particolare modo, negli emendamenti della Lega. È sempre pericoloso fare citazioni evangeliche prese a sé stanti, ma ricordo, anche in termini di realismo cristiano, quello che dice il paragrafo 298 del compendio della dottrina sociale della Chiesa: «La regolamentazione dei flussi migratori secondo criteri di equità e di equilibrio è una delle condizioni indispensabili per ottenere che gli inserimenti avvengano con le garanzie richieste dalla dignità della persona umana. Gli immigrati devono essere accolti in quanto persone e aiutati, insieme alle loro famiglie, ad integrarsi nella vita sociale. In tale prospettiva va rispettato e promosso il diritto al ricongiungimento familiare». Ecco, se sostenete questi emendamenti, se sostenete queste norme che limitano il diritto di contrarre matrimonio, che limitano il diritto di indossare abiti che segnalano la propria religione con pericolose tendenze a una limitazione dei diritti personali, non fate poi la retorica delle radici cristiane dell'Europa perché, oltre che violare la Costituzione, violate questi principi che ci provengono da questa tradizione e di cui la Costituzione è una delle forme più elevate di secolarizzazione.

reca disposizioni in materia di sicurezza pubblica e contiene una normativa svariata, in parte assolutamente nuova e in parte innestata su leggi esistenti, con modifiche che in alcuni punti - bisogna riconoscerlo - rispondono alle sfide di evidenti criticità e ad oggettive esigenze sociali di ordine e giustizia e che pertanto sono da considerare condivisibili sotto il profilo della lotta al crimine, nella misura in cui non debordano da questo ben definito ambito. Il testo in esame, purtroppo, però, risulta viziato - e, si potrebbe aggiungere, intenzionalmente inquinato dall'impropria e illegittima intrusione di disposizioni di ben altra natura, portatrici di intolleranza e xenofobia, concernenti in particolare il fenomeno dell'immigrazione, sia regolare, sia illegale: una materia che non dovrebbe essere assimilabile alla codificazione dei delitti di pena applicabili a reati di gravità infinitamente maggiore, quali quelli commessi dalle mafie, che quasi quotidianamente soffocano, e qualche volta insanguinano, tante parti del Paese. Su questo aspetto, però, tornerò dopo, con una considerazione di carattere più generale. Il provvedimento in esame fa infatti parte del cosiddetto pacchetto sicurezza, emanato a maggio, che prevedeva un decreto-legge, che - com'è normale - è già passato all'esame di questa Camera, e un disegno di legge: un pacchetto completo, quindi. Il decreto-legge fu varato in fretta, tanto che addirittura lo si è già dovuto correggere con un altro decreto-legge: questo ci fa pensare fa pensare al significato dell'uso e dell'abuso della decretazione d'urgenza. Lo si è corretto per la parte che riguardava la presenza dei soldati ed il numero del contingente dei soldati sulle strade.

fatto non con quell'adeguata e coerente attenzione che sarebbe necessaria quando, usciti dalla fase della campagna elettorale, invece, si incide realmente sulla qualità della vita dei cittadini. Da ultimo, nel decreto-legge, venivano anticipati anche alcuni contenuti del disegno di legge: si creavano, cioè, le condizioni prodromiche perché questo potesse avvenire. Veniva introdotta come aggravante l'ipotesi dell'immigrazione clandestina e i centri di permanenza temporanea venivano trasformati nella loro denominazione - questo aspetto è paradossale, perché contenuto all'interno di un decreto-legge - in centri di identificazione e di espulsione. Devo dire che allora criticai molto l'uso del decreto-legge, in parte per gli aspetto cui ho appena accennato, ma anche per la carenza di quei requisiti di necessità, urgenza ed omogeneità della materia che dovrebbero essere elementi fondamentali

Questi, più che badare alla sostanza, intesa come effettività e come possibilità di raggiungere il risultato, come attenzione - tante volte proclamata all'interno di quest'Aula alla qualità della vita dei cittadini, sembravano invece dare più peso all'impatto che questa norma avrebbe potuto produrre, nel suo effetto annuncio, soprattutto sulle popolazioni del Nord Italia, con

Non solo si prescinde dalla sostanza, ma si cerca di fatto di creare una specie di circolo vizioso in cui prima si alimenta la paura, spesso si strumentalizzano i dati che riguardano la

spazio si va ad annidare l'insicurezza potenziale dei cittadini e il peggioramento conseguente della qualità della vita degli stessi. In questo alternarsi tra paura e speranza si apre un baratro che finirà per allontanare i cittadini dalle istituzioni, perché si creerà un meccanismo di aspettativa a cui non saremo in grado di venire incontro e alla fine rischieremo di perdere veramente tutti.

Troviamo una sola norma che rappresenti un'inversione di tendenza rispetto al DPEF, in cui è prevista la diminuzione di 8.000 uomini nell'arco di tre anni? Troviamo una sola norma che dia il senso della possibilità di aumentare la capacità di intervento delle forze dell'ordine sul territorio? dell'ordine sul territorio? No, non c'è assolutamente nulla, ma c'è la capacità di impattare sull'esterno il fatto che ci si occupa dei cittadini del Nord.

su proposta del mio Gruppo), specialmente in materia di criminalità organizzata, di tutela penale rafforzata nei confronti di donne e minori stranieri vittime di sfruttamento e dell'immigrazione clandestina, e altre norme riprese dall'articolato dei quattro disegni di legge presentati nella scorsa legislatura

disposizioni di dubbia legittimità costituzionale, che però colpiscono e fanno rumore; il rischio tuttavia è che facciano molto più rumore nelle chiacchiere da bar che non all'interno delle aule dei tribunali.

Di cosa si tratta? Si tratta di assecondare le paure più ingiustificate ed eccessive, i pregiudizi più vieti e incivili? Si tratta di dare in testa all'immigrato, al diverso di lingua e cultura, ai più sfortunati, deboli e diseredati? Si tratta di questo? Con quale criterio, con quale logica - dobbiamo infatti chiederci - si affastellano nello stesso testo di legge, si gettano come in un frullatore, elementi fra i più disparati ed eterogenei, estranei gli uni agli altri, quali il delitto di mafia e il diritto al matrimonio dell'immigrato, i guadagni della criminalità organizzata e il permesso di soggiorno a punteggio per lo straniero, la condanna del criminale incallito e l'espulsione dell'innocuo clandestino o minore straniero già vittimizzato dai nuovi schiavisti, la videosorveglianza dei luoghi pubblici e il test di lingua italiana o la stipula di un accordo di integrazione per il permesso di soggiorno dello straniero? Non potevano, non potrebbero ancora, gli elementi attinenti all'ambito dell'immigrazione e della cittadinanza costituire un dispositivo a sé stante, venire stralciati da questo farraginoso disegno di legge dove c'entrano solo per rispondere ad esigenze, come dicevo prima, di immagine? Un disegno di legge che, come recita il titolo ufficiale, dovrebbe essenzialmente garantire la sicurezza pubblica dagli attacchi della micro e macrocriminalità. Ce lo possiamo o no dire che ciò cui bisognerebbe porre mano, come diceva giustamente la collega Adamo, è la legge Bossi-Fini, quella stessa legge

Cosa ha a che fare la repressione di elementari diritti umani degli immigrati, regolari e clandestini, con la repressione della criminalità organizzata? Assolutamente nulla. Ed è tale distorsione della realtà e della verità, tale forzatura, tale violenza al comune buon senso ed alle migliori regole della civiltà giuridica, paradosso dell'improprio connubio fra immigrazione e criminalità, Ma un criterio, una logica e una strategia in questo guazzabuglio concettuale di criminalità e immigrazione sono ravvisabili. Purtroppo, ci sono. Sono il criterio, la logica e la strategia del pregiudizio; il disegno politico di accostare, fino ad identificare, l'immagine dell'immigrato, dello straniero, con l'immagine del criminale, del nemico.

Randazzo - per esperienza diretta sulla loro pelle, le prove e i traumi, prima dello sradicamento e poi del riadattamento, prima dell'emigrazione e poi dell'immigrazione, le gioie dell'accettazione e della solidarietà e i dolori del rigetto, le vittorie e le sconfitte del multiculturalismo in distanti angoli della terra, solo costoro possono capire quanta insensibilità e, sotto certi aspetti, anche quanta disumanità vi sia in alcune delle nuove norme sull'immigrazione contenute in questo disegno di legge, ai cui punti salienti accenno molto brevemente. Penso al test di lingua italiana per l'accettazione formale e definitiva dei nuovi arrivati. Quanti milioni di italiani, di ogni epoca, di ogni età, di ogni condizione sociale e di ogni grado di scolarizzazione o di analfabetismo, che hanno raggiunto svariati livelli di prosperità sotto i cieli stranieri sarebbero stati respinti se i grandi Paesi d'immigrazione che li hanno ospitati avessero imposto loro l'obbligo della conoscenza preventiva delle lingue locali?

a punti, che possono conquistare come voti scolastici fino alla lode e al premio, oppure perdere fino al castigo e all'espulsione; al contempo, si ipotizza l'astrusa norma di un contratto d'integrazione come condizione del permesso di soggiorno. C'è ancora il reato di immigrazione clandestina di cui il relatore ha lamentato la derubricazione da delitto da codice penale a contravvenzione punibile con ammenda da cinquemila a diecimila euro. Ma non poteva che essere così. I motivi sono stati spiegati nei vari interventi in Commissione. Diversamente sarebbe stata soltanto la paralisi del sistema giudiziario e delle carceri. Altre violazioni di diritti umani e di norme internazionali, e persino di princìpi sanciti dalla nostra Costituzione, si ravvisano nell'estensione del termine massimo di detenzione, perché di questo si tratta, dello straniero nei centri di identificazione ed espulsione dagli attuali 60 giorni a 18 mesi, snaturando contemporaneamente e creando le condizioni per un ruolo diverso dei vecchi centri di permanenza temporanea, e soprattutto - permettetemi - nella subordinazione del diritto di matrimonio, che fa parte delle libertà fondamentali degli esseri umani, alla cittadinanza. ancora a tutto questo si aggiungono le discriminanti disposizioni per un registro dei senza fissa dimora, per l'istituzione di ronde civiche, di vigilantes, s'intuisce perfettamente che nelle categorie più deboli, indifese ed emarginate della società che si vogliono in particolare colpire ci sono proprio al primo posto, fra i più esposti e vulnerabili, tanti immigrati, l'anello debole della catena di un ordine razziale ancora da purificare secondo i canoni di una certa teologia pagana e padana. Sia chiaro a tutti che nulla al mondo, nessuna legge, anche la più draconiana, nessuno sbarramento di cemento o filo spinato, nessuna potenza navale, potrà bloccare il fenomeno degli arrivi dei clandestini, perché ci sarà sempre una parte di sventurati che un varco lo troverà ad ogni costo, anche a costo della vita, come avviene in quella tomba d'acqua che è diventato ormai il Canale di Sicilia. Il rischio della morte non può far paura a chi ogni giorno contempla con i propri occhi la morte dalla fame o dalla guerra o dal genocidio. Se non si apre la porta a chi bussa, chi bussa avrà la tentazione o la necessità di sfondare la porta. Con questa legge, impietosa, voluta ed imposta soprattutto dalla Lega Nord, ci troviamo di fronte ad una prospettiva di discriminazione istituzionalizzata elevata a sistema, l'ipocrisia senza fine! In un'Italia che continua a definirsi solidale e cristiana, dove molti dei politici promotori di questo disegno di legge quando ne hanno convenienza si ergono a paladini dei valori della Chiesa, la macabra realtà è che non si ha vergogna a difendere e diffondere una guerra alle minoranze. Sono questi i motivi che ci devono indurre ad una profonda riflessione, che ci portano a mettere a verbale queste considerazioni, sperando che un giorno non si possano e non si debbano realizzare e non si debba affermare: lo avevamo detto! detto! Penso che, alla luce di tutto questo, l'unica amara considerazione conclusiva è che all'atto della sua probabile approvazione il disegno di legge n. 733 sarà una legge da farci arrossire, agli occhi dell'Europa e del resto del mondo civile, senza contribuire significativamente a risolvere i reali problemi collegati alla sicurezza dei cittadini italiani.

Signor Presidente, il Gruppo dell'Italia dei Valori condivide molte norme del testo proposto dalle Commissioni. Infatti, come è stato ricordato anche dal presidente Vizzini, il disegno di legge governativo ha ripreso in molte parti i contenuti dei disegni di legge nn.

condividiamo; ciò che sicuramente manca a questo provvedimento è il completamento. Ossia, nel momento in cui si interviene modificando norme, inasprendo sanzioni, inserendo nuovi tipi di reati, ancor più marcato appare il vuoto, che tuttora persiste,

Parliamo di sicurezza, di necessità di rispondere alle esigenze dei cittadini secondo le nostre diverse angolazioni e prospettazioni - è chiaro che ognuno di noi può avere proprie convinzioni ma ciò che manca e che ci accomuna nel giudizio è che tutto quello che andiamo a fare cade in un settore malato della giustizia, quello del processo: il grande malato del sistema.

che i punti deboli della lotta alla mafia, che sicuramente esistono, sono i punti deboli di tutto il sistema; per una strana correlazione, infatti, l'azione antimafia viene bloccata dalla lentezza dei processi. Egli si chiedeva anche, nel documento depositato come si concilia l'esigenza di accelerare il corso della giustizia con la circolare del Ministero della giustizia che invita comunque a ridurre le spese ed a far funzionare al minimo gli uffici. Questo è quanto scritto nel documento che ci è stato consegnato. Su questo fronte c'è un totale vuoto. Continuiamo a muoverci nella direzione dell'inasprimento, intervenendo sulla parte sostanziale del diritto, del diritto, e ad essere totalmente assenti sulla parte processuale, cioè sulla macchina che poi deve consentire la celebrazione dei processi, l'effettività della pena e l'ineluttabilità delle decisioni. Quando nella scorsa legislatura i cui testi in questa materia sono stati ripresi anche dal Governo - affrontammo tale problema lo facemmo nella contestualità della proposta di riforma dei codici.

si mosse prospettando soluzioni processuali che riguardavano la possibilità di celebrare i processi. La fine della legislatura ha impedito questo percorso, ma era una visione di insieme, era armonica: si interveniva sul piano sostanziale e sul piano processuale. Invece ciò cui noi stiamo assistendo è che si interviene dal punto di vista sostanziale inasprendo le pene o individuando nuovi reati, però non si interviene sul processo. Si tagliano le risorse (e vale sempre ricordare che, nell'arco di un triennio, le risorse per la giustizia verranno defalcate del 40,5

perché questo è un provvedimento che contiene una norma di mera propaganda. Con l'articolo 19 si introduce il reato di ingresso e di permanenza irregolare

con applicazione in riferimento specifico alla normativa del giudice di pace. Pensate veramente che l'immigrato irregolare paghi l'ammenda di 5.000 euro? Non credo che voi lo pensiate, anche perché sapete benissimo che il giudice di pace, nel momento in cui il condannato è insolvente, può e deve applicare altri tipi di pene. Quali sono le altre pene che dovrà applicare?

Il giudice di pace che cosa potrà fare? Qualora il condannato lo richieda,

che occorre aprire una posizione assicurativa, previdenziale e assistenziale. Quindi, questa soluzione è impraticabile. Allora, il giudice di pace dovrà convertire la pena pecuniaria con l'obbligo di permanenza domiciliare

perché prevedendo la punizione sia dell'irregolare che fa ingresso (reato istantaneo), sia dell'irregolare che si trattiene nel nostro Paese (reato permanente), fermo il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, la platea dei destinatari dei processi è costituita da centinaia di migliaia di persone, vale a dire che tutti gli irregolari nel nostro Paese devono essere processati.

inoltre, un costo di 650 euro a testa per il gratuito patrocinio. Moltiplicando 650 euro - calcolo effettuato dal Ministero nella scheda tecnica allegata al disegno di legge - per centinaia di migliaia di posizioni,

c'era bisogno di mettere in moto questa macchina giudiziaria, già in affanno, appesantendola di centinaia di migliaia di processi, con un esborso di alcune centinaia di milioni; a quale risultato

si poteva e si può arrivare ad applicare l'espulsione amministrativa, che è disposta proprio nel caso in cui lo straniero è entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera e non è stato respinto.

per il sistema giustizia in affanno, celebrando processi inutili con sanzioni inutili e con costi enormi?

aspetti concreti perché l'espulsione amministrativa è già prevista dal nostro sistema e ha già superato il vaglio di costituzionalità con una sentenza della Corte costituzionale del 2004: perché non applicate quella norma? La difficoltà di applicazione della norma non viene risolta dal passaggio attraverso la celebrazione di centinaia di migliaia di processi. L'altra norma che rappresenta sicuramente qualcosa di veramente grave è l'inserimento,

previo parere del comitato provinciale (non è un parere vincolante, è un semplice parere), sono legittimati ad avvalersi

non ai fini della denunzia. Presidente Vizzini, quando lei dice che dobbiamo scegliere tra l'omertà e la collaborazione, lei usa un'espressione un po' propagandistica. Il cittadino può denunziare quando vuole i reati; questa norma non ha una funzione pedagogica, nel senso che non si sta dicendo ai cittadini di denunziare i reati. Si sta dicendo che gli enti locali possono avvalersi delle associazioni di cittadini per cooperare nello svolgimento dell'attività di presidio del territorio, cioè di un'attività che devono svolgere le forze di polizia. Presidio del territorio vuol dire presenza sul territorio. E come lo faranno? Armati? Presidio del territorio per contrastare la criminalità significa anche potersi difendere dall'attacco di un criminale e quindi, anche al solo scopo difensivo, si dovrà consentire che le associazioni di cittadini che devono presidiare il territorio possano essere armate. Anche a scopi difensivi. Ma cosa stiamo facendo nel nostro Paese? Veramente stiamo perdendo il senso della misura? Noi stiamo introducendo una polizia parallela, affidata agli enti locali, che dovranno munirsi di un parere non vincolante e che potranno, a titolo oneroso (non c'è scritto a titolo gratuito), avvalersi di associazioni tra cittadini. Li pagheranno e faranno svolgere loro un servizio di polizia che spetta invece allo Stato, che è un compito primario dello Stato, al quale noi non intendiamo rinunziare, perché appartiene ai principi dello Stato di diritto. La sicurezza pubblica e l'ordine pubblico sono compito dello Stato,

vedere lo Stato come titolare di determinati poteri e non sottrarre allo Stato questi poteri, ma al contrario potenziare lo Stato nell'esercizio del suo potere, per la tutela e la sicurezza dei cittadini. Voi state così rinunziando a qualcosa che dovrebbe far parte della cultura, anche politica, di una parte di questa maggioranza. Io rimango veramente sorpreso di come si possa, attraverso questa ulteriore norma manifesto, chiaramente incostituzionale, prospettare e far pensare agli italiani che abbiamo risolto il problema dell'ordine pubblico, perché ogni Comune potrà munirsi di gruppi di volontari che potranno girare la notte armati per tutelare la tranquillità dei cittadini che sono nelle loro case, sottraendo alla polizia quello che è il compito primario della polizia

questo disegno di legge assolutamente una norma manifesto, contraria allo spirito che dovrebbe animare chi pone al centro degli interessi la tutela del cittadino, la propria sicurezza e il contrasto al crimine.

originario del disegno di legge in esame è dedicato ad un aspetto della sicurezza molto specifico: quello, ahimè, della sicurezza stradale. Dico ahimè perché i dati allarmanti circa la mortalità sulle strade, nonché i troppi frequenti fatti di cronaca che, soprattutto il lunedì, ci impongono il triste rito della conta dei morti e feriti del weekend hanno imposto un giusto e opportuno intervento nel senso dell'inasprimento delle sanzioni per chi viene sorpreso alla guida in stato di ebbrezza. Proprio questo aspetto così specifico della sicurezza, come più in generale trattata nel testo legislativo, ci rimanda ad un fenomeno molto diffuso, ma purtroppo sottovalutato: quello dell'uso e dell'abuso di sostanze alcoliche, ma non solo. Signor Presidente, onorevoli colleghi, alcuni dati devono farci riflettere sulla dimensione più generale di questa che rappresenta una vera e propria emergenza, non solo sociale ma anche sanitaria. Ogni anno nell'Unione europea 195.000 persone muoiono per cause riconducibili all'alcol. Una recente stima, condotta per l'Italia con metodologie adottate dall'OMS, indica in 24.000 il numero delle morti annuali causate dall'alcol fra i soggetti in età superiore ai 20 anni, 7.000 delle quali riguardano le sole donne. Secondo dati ISTAT, nel 2006 si sono verificati più di 6.000 incidenti stradali causati dallo stato psicofisico alterato del conducente; di questi il 71 per cento, pari a più di 4.200 casi, è stato causato da guida in stato di ebbrezza da alcol e da altre droghe. È sulla base di questi dati, a mio avviso particolarmente preoccupanti, che voglio sviluppare una serie di considerazioni e raccomandazioni, che rivolgo al Governo, volte a rendere ancora più efficace il provvedimento legislativo in discussione. Infatti, signor Presidente, il semplice inasprimento delle sanzioni previsto per chi viene sorpreso a guidare sotto l'effetto dell'alcol potrebbe indurre a ritenere che questa drammatica emergenza sociale possa essere risolta solo attraverso la criminalizzazione della sostanza o, peggio ancora, dei suoi consumatori. Questi, in realtà, costituiscono una categoria estremamente eterogenea di persone nella quale possiamo e dobbiamo riconoscere chi fa un uso moderato dell'alcool, chi ne abusa occasionalmente e chi è affetto da una vera e propria dipendenza. Ne consegue che l'accertamento, pur non prescindendo dall'applicazione della sanzione, può diventare l'occasione per un'operazione di informazione e di maggiore sensibilizzazione verso il problema degli effetti dell'alcol alla guida dell'automezzo. Nel caso della dipendenza e/o uso patologico dell'alcol, la sanzione può e deve essere accompagnata dall'avvio di un intervento terapeutico e riabilitativo, se vuole essere veramente efficace. Questo consentirà, a medio termine, una maggiore sicurezza sociale, un risparmio di vite umane e, naturalmente, di risorse economiche per effetto degli interventi di prevenzione delle recidive, su cui la semplice sanzione non ha alcun effetto. E questo è un dato che è stato dimostrato nel tempo. Signor Presidente, onorevoli colleghi, è bene riconoscere nel soggetto alcol-dipendente, laddove individuato, l'esistenza di un vero e proprio disturbo che travalica il vero ambito sociale per interessare anche quello clinico e riabilitativo. Il soggetto che abitualmente abusa di sostanze alcoliche non è, troppo semplicisticamente, affetto da un vizio, ma da una malattia dalle complesse sfaccettature cliniche. L'abuso di alcol rappresenta oggi una vera e propria emergenza sociale, destinata ad aggravarsi se non si avvia subito un processo di ricollocazione del problema anche all'interno di una prospettiva clinico-terapeutica che, come tale, deve essere caratterizzata da opportuni percorsi di cura, riabilitazione e reinserimento. In conclusione, cari colleghi, il tema della sicurezza non può non tener conto delle strategiche necessità che questi fenomeni emergenziali impongono. L'alcolismo e le tossicodipendenze debbono rappresentare un momento qualificante dell'agenda del Governo, integrando gli interventi sanzionatori con un coinvolgimento in rete di varie istituzioni, quali università, servizi ospedalieri e servizi territoriali. Questo allo scopo, in prima istanza, di individuare e gestire strategie preventive che possano così diventare appropriatamente efficaci. Cerchiamo, cari colleghi, di non colpevolizzare tutti quelli che occasionalmente, a cena, vogliono assaporare un buon bicchiere di vino italiano.

tutti condividono il principio che la sicurezza dei cittadini e di tutti coloro che vivono o visitano il nostro Paese, a qualsiasi titolo lo facciano, è un bene primario, da assicurare e custodire. Ma su come questo bene primario venga conseguito e rafforzato le opinioni divergono. Per quanto riguarda il disegno di legge in esame, specialmente nella parte attinente all'immigrazione, le divergenze sono ampie e profonde, perché il testo voluto dalla maggioranza contiene norme in alcuni casi inefficaci, in altri lesive dei diritti individuali, in altri ancora intrusive nella normale vita di italiani e stranieri. Sotto il falso pretesto di frenare l'irregolarità - un principio sul quale, in astratto, tutti sono d'accordo - passa invece una sola logica: rendere difficile la vita agli immigrati, europei e non europei, regolari e irregolari e, in qualche caso, anche agli italiani. Già il decreto-legge approvato nel luglio scorso conteneva il chiaro annuncio: l'aggravante della pena pari ad un terzo per i reati compiuti dall'immigrato irregolare, anche per colui - per intendersi - cui fosse scaduto il permesso di soggiorno il giorno prima. Una norma iniqua, che considera l'irregolarità come un'aggravante comune, come l'avere agito per abietti motivi o con crudeltà. Sotto la pressione della Comunità europea, poi, il Ministro dell'interno ha dovuto ritirare un decreto legislativo che imponeva forti restrizioni alla libera circolazione dei cittadini europei, mediante l'allontanamento di chi fosse sprovvisto di adeguati requisiti di reddito. Una disposizione chiaramente contraria ai princìpi comunitari della libera circolazione nello spazio europeo. Sulla questione dei rom e della loro schedatura-censimento, purtroppo avvenuta all'ombra della Croce Rossa, solo alcune acrobazie hanno impedito le censure comunitarie, ma non certo quelle dell'opinione pubblica e di molte istituzioni internazionali. La mozione approvata alla Camera sulle cosiddette classi ponte, o differenziate, mostra poi il chiaro intento di orientare la politica scolastica verso la segmentazione, anziché verso la comunanza, degli allievi a seconda dell'origine etnico-linguistica. Con il disegno di legge in questione, la maggioranza, ostaggio della Lega, sta facendo di peggio. Non illuda il fatto che il Governo abbia innestato una clamorosa marcia indietro sul reato di immigrazione clandestina, che avrebbe comportato l'arresto, il processo, l'espulsione di tutti gli irregolari, comprese le centinaia di migliaia di collaboratrici familiari. Una norma tanto proterva quanto inattuabile e ritirata più per la sua manifesta dannosità e impraticabilità (sistema carcerario che scoppia, tribunali intasati, costo delle espulsioni) che per le diffuse proteste dell'opinione pubblica, laica e religiosa. Con la nuova formulazione dell'articolo 9, l'irregolarità continua ad essere un reato, derubricato da delitto a contravvenzione, ed è punibile con un'ammenda. La denuncia comporta l'espulsione; se questa è eseguita, il giudice dichiara non esservi luogo a procedere. Questa formulazione più blanda - che ha aspetti giuridici assai controversi - non eviterà l'intasamento degli uffici giudiziari né le difficoltà logistiche per decine o centinaia di migliaia di espulsioni. Occorre ricordare che il numero degli irregolari sul nostro territorio è sconosciuto e variamente indicato da fonti responsabili in cifre comprese tra mezzo milione e un milione. Una massa di individui - quasi tutti operose lavoratrici e lavoratori - la cui sorte non può essere regolata da espulsioni di massa. Occorre poi segnalare che il Governo non tiene conto delle indicazioni della direttiva europea, in corso di approvazione, che prevede che all'immigrato irregolare che non sia un pericolo per la sicurezza e l'ordine pubblico (cioè la stragrande maggioranza) debba essere concesso un periodo compreso tra i sette e i trenta giorni per ottemperare volontariamente all'ordine di rimpatrio, periodo prorogabile in circostanze particolari quali l'esistenza di figli a scuola, i legami familiari, la durata del soggiorno. Il fatto è che l'irregolarità affonda le radici nelle vaste dimensioni dell'economia sommersa e si alimenta per le regole di ammissione contenute nella legge Bossi-Fini che rendono difficile l'ingresso legale all'immigrato che cerca un posto di lavoro, anche quando il posto esiste: solo prosciugando la prima e riformando le seconde si può pensare di riportare a maggiore legalità l'immigrazione. Si dirà che sono politiche troppo impegnative perché l'attuale Governo le voglia perseguire; oppure che un certo elettorato non vuole sentir parlare di sconfessione della Bossi-Fini (anche se ha sortito effetti disastrosi). Eppure si tratterebbe solo di prendere atto con realismo della realtà, e cioè che il datore di lavoro artigiano o piccolo imprenditore o famiglia non è attrezzato per reperire all'estero, alla cieca, senza un incontro effettivo, il lavoratore che necessita. Così la legge viene aggirata: si arriva regolarmente, si cerca lavoro, si trova e si entra nell'irregolarità. È questa la ragione per la quale il serbatoio dell'irregolarità continua ad alimentarsi, ed a richiedere - stando alla lettera delle legge - un numero crescente di espulsioni. Ma il Governo è anche sordo nei riguardi di altre proposte di buon senso quale quella, per esempio, di incentivare il ritorno volontario dell'irregolare, evitando quello coatto, che è molto costoso e che dovrebbe essere l'eccezione e non la regola. Oppure quella di dare permessi di soggiorno premiali agli irregolari che abbiano un lavoro, o che lo ricerchino, o che abbiano legami familiari, o siano da tempo nel nostro Paese e bene inseriti nella società, caratteristiche proprie di larga parte dei migranti non in regola oggi presenti in Italia. Il florilegio delle misure che tendono a restringere i diritti e a disseminare difficoltà nella vita degli immigrati, come in quella degli italiani, è ampio e variato. Non ho tempo per passarlo in rassegna e mi limito a cogliere i fiori più amari. Non era passato in Commissione l'emendamento della Lega che tendeva a limitare l'accesso alle cure sanitarie degli irregolari, con gravi pericoli per la sanità pubblica, (ma poi è stato ripresentato qui in Aula), ma è passata la norma che autorizza gli enti locali ad avvalersi di ronde di cittadini per cooperare nell'attività di presidio del territorio, con un'inaccettabile intrusione del privato nel mantenimento dell'ordine pubblico. Uno strumento che, se manovrato irresponsabilmente, può creare gravissimi problemi di conflitto sociale. Si istituisce presso il Ministero dell'interno un registro dei senza fissa dimora italiani e stranieri le cui finalità non sono precisate, ma che suona minaccioso come le ronde e che rischia di bollare con un marchio assurdo individui in gravi condizioni di disagio, debolezza e vulnerabilità, col rischio di cadere nel ridicolo (sì, nel ridicolo): si può essere senza fissa dimora oggi e non domani; si può esserlo in un Comune e non in un altro. Chi e come e con quali criteri curerà l'iscrizione e la cancellazione dal registro? E, soprattutto, a che serve il registro? Si burocratizza la spedizione di denaro all'estero mediante *money transfer*, veicolo semplice e poco costoso per trasferire le rimesse, col rischio di deviarle verso canali illegali e più rischiosi. Effetti devastanti - mi soffermo velocemente su questo aspetto - avrà poi sulla tenuta delle anagrafi (che sono uno strumento essenziale di governo e di amministrazione, la base per le liste elettorali, il fondamento delle rilevazioni e delle indagini statistiche) la norma che subordina l'iscrizione anagrafica (vuoi per lo straniero regolare, vuoi per l'italiano) alla verifica dell'idoneità sanitaria dell'abitazione. In linea di diritto questa norma potrebbe portare alla cancellazione dalle anagrafi di milioni di famiglie che vivono in abitazioni degradate e antigieniche. Essa renderebbe insicura e incompleta l'iscrizione degli stranieri regolari in anagrafe, atto che determina l'ingresso nel sistema statistico informativo della popolazione. La norma potrebbe essere facilmente aggirata segnalando abitazioni di comodo come residenza. È una norma che sarebbe sicuramente interpretata in maniera diseguale sul territorio, alterando il grado di completezza e di copertura dell'anagrafe. Essa, infine, non è a costo zero: agli uffici di anagrafe non spetta per legge la verifica delle condizioni delle abitazioni; altri uffici tecnici dovrebbe eseguirla, con costi elevatissimi. Con un'altra norma si impedisce il matrimonio (diritto umano fondamentale) all'irregolare (così come facevano alcuni padroni di schiavi nelle piantagioni). Al regolare si preclude la carta di lungo-soggiornante (si badi: non il diritto di voto o la cittadinanza) se non viene superato un esame di italiano. Si propone un permesso di soggiorno a punti legato al processo di integrazione, del quale non vengono precisate né le tappe, né le modalità, né i contenuti. Al rinnovo del permesso, per chi non ha compiuto il percorso assegnato (a giudizio discrezionale delle autorità) si procede all'espulsione. Se non fossimo sbalorditi dal contenuto di questa norma improvvisata, saremmo curiosi di sapere in che modo si pensi di attuarla. Si introduce una tassa di 200 euro per ogni permesso di soggiorno concesso o rinnovato: un balzello odioso e pesante, la cui destinazione non è specificata. Almeno fosse indirizzato, questo prelievo, a rendere efficaci e veloci le procedure di rilascio e rinnovo dei permessi. Quanto sopra ho detto tiene conto del testo proposto dalle Commissioni 1a e 2a, ma non degli ulteriori emendamenti presentati in Aula, tra i quali si distinguono quelli della Lega, espressione delle posizioni più retrive e più miopi in tema di immigrazione. L'idea di far pagare agli irregolari gli interventi di pronto soccorso e di comunicare l'identità di chi non può farlo alle autorità di pubblica sicurezza è contraria ad ogni principio umanitario. Essa può venire in mente solo ad un movimento politico che - quando fa comodo invoca la strenua difesa dei principi della dottrina cristiana e cattolica, ma che, nella versione "padanica" (non dico nemmeno padania) su temi migratori, è rappresentata dalla croce celtica più che dalla croce di Cristo. Il blocco di due anni dell'immigrazione non sta in piedi per mille e una ragione: la crisi morderà in alcune attività, ma non in altre; i ricongiungimenti familiari non potranno essere sospesi e via enumerando; assai meglio sarebbe prolungare da sei mesi a dodici la validità del permesso di soggiorno per ricerca di un nuovo lavoro ed evitare che la crisi non spinga immediatamente nell'illegalità i lavoratori stranieri che restano disoccupati. La realtà è, cari colleghi della maggioranza, che non esprimete una politica dell'immigrazione - il fenomeno sociale più rilevante di questo inizio di secolo - e affidate la soluzione di ogni problema ad una normativa che impone solo divieti, controlli, limitazioni, come quella contenuta nei vari involucri incartati nel pacchetto sicurezza, il vostro regalo di Natale per gli immigrati. È un regalo che contiene un messaggio articolato in disposizioni inattuabili, con formulazioni pasticciate, e condito dal disprezzo dei diritti umani, con un chiaro avvertimento: la vita dell'immigrato sia difficile, la sua cacciata facile.

mi permettono di prendermi una libertà e di intervenire più sul contesto e sulla filosofia di questo provvedimento. Il contesto, che è

Non c'è ovviamente un rapporto diretto tra la costruzione della paura e l'ossatura giuridica del provvedimento che stiamo esaminando, però, c'è una relazione larga. Queste leggi vengono fuori perché in Italia c'è chi ha i mezzi, la voglia, la potenza per esercitare tale propaganda profonda, pervasiva, che entra in tutte le case e che ripete con monotona serietà e continua capacità intimidatoria questa realtà plumbea: l'Italia versa in una situazione in cui la criminalità non è più sotto controllo, dobbiamo temere ed essere paurosi. La cosa curiosa e il risvolto ironico di questa faccenda sono che la potenza del mezzo propagandistico talvolta si esercita a rovescio. Ricordo, ad esempio, che durante il primo Governo Berlusconi vi fu un momento di involontaria ironia, in cui

cento. Si potevano immaginare, cioè, senza fatica gli italiani che emigravano verso l'Albania, perché il rapporto ormai era completamente rovesciato grazie alle virtù salvifiche del Governo. Dunque, la paura. Dall'imposizione della paura nasce qualcosa che alcuni esperti di diritto hanno definito populismo penale. Luigi Ferrajoli, grande giurista dei nostri giorni, che ha appena licenziato tre volumi di «*Principia iuris*», ricorda in un suo scritto questa espressione, attribuita a Denis Salas e Eduardo Jorge Prats. Che cosa è il populismo penale? È il modo per ottenere per via demagogica - cito testualmente - il consenso popolare rispondendo alla paura generata nella popolazione dalla criminalità di strada. di strada. Ma non c'è solo la paura, c'è l'immanenza della propaganda della paura, perché forse, se ci fosse solo la criminalità di strada, non basterebbe. Dunque, il populismo penale si configura come una sorta di uso congiunturale del diritto penale, che va direttamente in senso soltanto repressivo, antigarantista e, oltretutto, nella sua essenza appare inefficace a promuovere davvero la prevenzione del crimine. Siamo nel regno della tolleranza zero

attraversando i mari e gli oceani, dilagando con una formula, anche questa, di salvezza. La tolleranza zero è, nella sua stringatezza, un'utopia reazionaria: è l'idea che si possano eliminare i delitti, e questa possibilità di eliminare il delitto presuppone un'involuzione totalitaria del sistema politico.

articolato la sua trattazione basandosi nell'analisi della storia giuridica e penale dell'Europa sulla diffusione del *panopticum*, un tipo di prigione dove il secondino, il controllore, dal centro di uno spazio circolare può sorvegliare in tutte le direzioni della rosa dei venti i vari bracci

La tolleranza zero si accoppia ad una sorta di visione di un *panopticum* mondiale, un *panopticum* sociale, quest'idea che si possa sorvegliare e punire in tutte le direzioni. La tolleranza zero è vacua, perché naufraga, si interrompe contro qualsiasi evento che la mette in discussione. Il crimine di per sé non è eliminabile; il delitto di per sé non è eliminabile, nemmeno con la tolleranza zero, nemmeno con il *panopticum*. Anzi, un eccesso di attenzione repressiva può essere addirittura il meccanismo che scatena un vieppiù, una crescita della possibilità di crimine.

totale. Si assiste, infatti, con una certa facilità, ad una sorta di duplicazione del diritto penale; un diritto penale che, da una parte, si configura come esercizio della legge potente nei confronti - in generale - dei deboli o dei prepotenti di basso grado sociale oppure degli immigrati, degli estranei e dei nemici

con una forza sempre più stringente e con un'intenzione sempre più repressiva, a chi non si può difendere e a chi spesso non ha nemmeno compiuto reati, ma è solo colpevole di una condizione.

l'attore di una condizione spesso involontaria. Ciò determina, nel concreto, fenomeni repellenti di esposizione alla violenza omicida. Non ritorno su fatti noti, ma abbiamo avuto casi simili ai linciaggi di un tempo,

ma ci sono anche i cittadini che da sé prendono l'iniziativa. Questi sono fenomeni terribili. Abbiamo creato una situazione in cui il cittadino, a un certo punto, si arroga il diritto di essere esso stesso l'attore della legge, di farsi legge e determinare una situazione per cui si può andare ad incendiare

di organi di stampa, di vicini, di prossimi. Si tratta di un'atmosfera molto pericolosa, che mi fa giudicare ulteriormente più pericolosa l'idea che si possa ricorrere, nell'esercitare il controllo sociale su fenomeni che sono di per sé slabbrati, magmatici e policentrici, alle ronde. Queste ultime sono un fenomeno di straordinario pericolo sociale.

una cosa che ci costringe quasi ad esagerare nella controproposta. Dobbiamo guardare a questi fenomeni non pensando alla alla prevenzione come l'esercizio di un'azione penale. La vera prevenzione, voglio esagerare, è pre-penale. La vera prevenzione viene prima di tutto il grande carico del grande macchinismo, dell'iniziativa giudiziaria, di polizia, e così via. La vera prevenzione è saper guardare con occhi sereni la realtà sociale, che non è poi così disastrosa, perché la situazione italiana è tutt'altro che catastrofica dal punto di vista dell'ordine sociale.

promozione di una solidarietà sociale. So bene che dire queste cose comporta l'accusa di indulgere in una sorta di retorica dolciastra (siamo troppo buoni, si pretende di esercitare la bontà coatta). Non penso che sia soltanto retorica dolciastra. Penso che nei confronti di queste dinamiche sociali di difficilissimo governo dovremmo recuperare quel senso di critica dell'individualismo esasperato. È piuttosto l'individualismo esasperato un'autentica modificazione della condizione umana. Nessuno di noi si è fatto da sé, neanche quelli che pensano di essere gli autori di se stessi. Noi siamo i figli, il frutto delle infinite persone che abbiano incontrato e che ci hanno influenzato, dei buoni e dei cattivi maestri, di chi ci ha insegnato qualcosa di importante e di chi invece ci ha fatto capire che si può anche insegnare in modo malvagio. E tuttavia questa è una relazione. Noi siamo i figli delle esperienze degli altri; siamo i figli dei libri che abbiamo letto e persino di quelli che non abbiamo letto, che sappiamo che esistono e a cui facciamo riferimento; siamo figli delle bibliografie e delle memorie degli altri uomini. Non si può pensare di esercitare un'azione sociale dimenticando questo fenomeno fondamentale della specie umana. Lévinas, un filosofo poco conosciuto, un omino piccolo piccolo, molto modesto, che nel dicembre del 1989 ricevette il premio Balzan per la filosofia a Berna,

o la donna? Si riconosce nel colloquio dei volti, nel fatto che un volto guarda l'altro volto, nel fatto che uno sguardo incontra un altro sguardo. Non c'è il solipsismo dell'uomo. L'uomo solipsista non esiste. È un dato che non c'è. La cosa fondamentale è questo incontro dell'altro, lo specchiarsi nell'altro, l'interrogarsi nell'altro. Penso che una legislazione capace di recuperare questo senso profondo dell'umanità potrebbe forse produrre delle leggi migliori.

Noi abbiamo utilizzato il nostro tempo e ci siamo. Meglio un ostruzionismo parlamentare serio, che nel caso di specie non c'è stato, che il menefreghismo della maggioranza, che sventola la bandiera di un disegno di legge in cui evidentemente non crede neppure lei.